Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di

dei deputati. Era prevista la commemorazione della ricorrenza dell'arrivo a Roma del Milite Ignoto partito da Aquileia cento anni fa, com'è noto, il Regolamento impone, subito dopo l'apposizione della fiducia, un silenzio tombale in Aula, per cui non posso neanche dare la parola al Presidente del Gruppo Fratelli d'Italia

darò comunque la parola a chi la chiederà sull'ordine dei lavori e troveremo anche il tempo per la commemorazione. Presidente Ciriani, le chiedo perdono per non poterle dare la parola, ma la sua contrarietà all'apposizione della fiducia è così evidente dall'applauso che forse ogni parola sarebbe superflua. La seduta è sospesa.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

posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. La discussione sulla fiducia, per la quale è stata attribuita un'ora in base a specifiche richieste dei Gruppi, avrà inizio al termine della commemorazione sul 100° anniversario della traslazione del Milite Ignoto. Seguiranno le

che affronteremo dopo e che appartiene alla polemica politica, anche molto giustificata a mio avviso. Il mio intervento è invece riferito a una ricorrenza che dovrebbe unire tutti. Mi spiace, visto che è stato preannunziato nella riunione dei Capigruppo, vedere largamente assenti molti parlamentari, soprattutto dell'emiciclo opposto al nostro. La ricorrenza a cui faccio riferimento

posizionate in maniera che non fosse possibile identificare la provenienza dei soldati che vi erano custoditi, soldati caduti nei luoghi simbolo nella Prima guerra mondiale, dove i nostri militari, contro un esercito che allora era il più forte del mondo, quello austro-ungarico, si erano distinti per valore, abnegazione e sacrificio fino alla morte, per ridare unità alla nostra Patria, per completare quel Risorgimento a cui tanti italiani avevano anelato. Era stato il governo Giolitti negli ultimi giorni della sua vita, prima che cadesse per una maggioranza troppo risicata, a deliberare, sempre nel 1921, che la salma di un soldato ignoto venisse custodita e sepolta sotto la dea Roma, in quello che da quel momento in poi si chiamerà l'Altare della Patria, che è il Vittoriano. Torniamo a quel 28 ottobre. Una madre, simbolo delle madri di tanti caduti, noti e soprattutto ignoti, che avevano dato la vita nelle trincee, ma anche nel mare e nei nei luoghi di battaglia, Maria Bergamas, sfilò davanti a quelle 11 bare, di cui non conosceva neanche la provenienza, certamente non il nome dei soldati caduti, e si fermò senza indecisioni di fronte a una di esse: fu quella la bara prescelta, una bara in metallo con all'interno il corpo di un soldato e all'esterno un elmetto, una bandiera tricolore e un fucile. Venne apposta su un affusto di cannone, tuttora custodito nel museo, e su un treno iniziò una marcia lenta e silenziosa che l'avrebbe portata fino a Roma. In quell'Italia dolente ma vittoriosa si manifestò qualcosa di mai più visto nella storia italiana: lungo il percorso di quel treno migliaia e migliaia di persone si accostarono ai binari in ginocchio, riconoscendo a quel Milite Ignoto gli onori che tutta l'Italia doveva e deve a chi si immolò per la Patria, per l'indipendenza, per la libertà e per l'unità della nostra Nazione. Maria Bergamas aveva un figlio, si chiamava Antonio; era caduto, era stato sepolto, ma poi, nel cimitero dove era stato sepolto, c'era stato un bombardamento, quindi era diventato impossibile riconoscere i singoli corpi. Maria Bergamas si accostò anche alle altre bare, che furono e sono tutt'ora sepolte nel cimitero vicino alla Basilica di Aquileia, ma la salma del Milite Ignoto che fu

rappresenta o dovrebbe rappresentare quell'amore dell'Italia per i propri figli, per la propria storia, per la propria cultura, per la propria libertà, per la propria indipendenza, per la propria sovranità. Al Milite Ignoto, Presidente, agli uomini e alle donne con le stellette che ancora oggi onorano la nostra Nazione, e che a mio avviso sono la migliore gioventù di questa Italia, va il nostro perdurante, totale amore e riconoscimento. *(Applausi)*. Signor Presidente, ho apprezzato molto l'intervento del senatore La Russa, specialmente per i toni (di solito è più focoso), magari è la ricorrenza di oggi. Faccio presente che, però, quando parla di assenza nell'emiciclo, forse non ha guardato davanti ai suoi banchi: saranno tutti fuori davanti al televisore; comunque sia, andiamo avanti. Oggi, 4 novembre, celebriamo il Milite Ignoto: un'espressione coniata in seguito al Primo conflitto mondiale per individuare tutti coloro che persero la vita in guerra senza mai essere identificati; la forma più solenne per indicare il sacrificio e la massima dedizione per il proprio Paese. Un passaggio fondamentale della nostra storia, lasciato in eredità a tutti noi e che rimarrà eterno anche per le future generazioni. Oggi sono passati cent'anni dal momento in cui si decise simbolicamente di tumulare al Vittoriano di Roma i resti di uno dei tanti, troppi nostri soldati caduti al fronte. Le spoglie del soldato privo di nome furono messe in cammino su un treno speciale, che prevedeva una sosta di qualche minuto in oltre 100 stazioni d'Italia. Un'iniziativa che suscitò grande commozione tra le folle, che si inginocchiavano al passaggio del treno immedesimandosi nel dolore straziante di un figlio o di una madre, riuscendo a unire l'intero Paese. Un messaggio di unità quanto mai attuale che resta scolpito nella nostra storia, immutato dinanzi al passare del tempo. Oggi, rispetto a un secolo fa, trovo molte similitudini: anche oggi, come allora, siamo di fronte a un'Italia da ricostruire, dopo aver superato un periodo terribile. Il Covid, infatti, può senz'altro essere paragonato a una guerra per il numero di vittime che in Italia ha recentemente superato la cifra di 132.000. Anche ai loro più cari affetti voglio dedicare oggi un commosso pensiero. Riguardo alla celebrazione odierna ritengo essenziale che vengano create molte più occasioni, soprattutto dedicate ai nostri giovani, per ricordare il passato più recente del nostro Paese; in primo luogo nelle scuole, dove ritengo sia fondamentale insegnare a tenere viva la memoria, perché oggi siamo ciò che siamo stati e domani saremo ciò che oggi siamo. Concludo, ricordando con estrema umiltà un nostro collega che nel 1950 fece parte - anche se per un brevissimo periodo - della prima legislatura: Carlo Alberto Salustri, il grande Trilussa, nominato senatore a vita dal presidente Luigi Einaudi. Con amara e macabra ironia, il poeta romano si definì senatore in morte; da tempo malato, mancò venti giorni dopo la nomina. Nel 1915 Trilussa compose «Fra cent'anni», e nella giornata di oggi, nel ricordo dei caduti e del Milite Ignoto, vale la pena andare a riscoprire quel testo e a goderselo tutto. Un testo che allego al mio intervento in modo che possa essere recepito nel Resoconto stenografico.

Sinteticamente terra dei padri, Patria, ha questo significato ed è quello che noi chiediamo. Chiediamo, appunto, di ricordare il sacrificio per la Patria, un sacrificio che chiede a un'ultima riflessione - soprattutto a noi come istituzione, non semplicemente il ricordo. Celebrare e commemorare sono parole molto importanti, ma assomigliano a chiacchiere vuote, se non ci sono i fatti.

ricordiamoci concretamente di proteggere lo scudo e la spada delle nostre libertà, del nostro vivere, della nostra identità: le Forze armate. E come possiamo farlo? Non solo con le parole, ma anche con i fatti, i provvedimenti e gli stanziamenti. e gli stanziamenti. Invito dunque tutti noi a difendere chi ci difende, a difendere chi protegge quei valori che a parole qui tutti condividiamo. Voglio quindi

L'invito è soprattutto a noi: sosteniamo concretamente le Forze armate e parliamo serenamente di stanziamenti per la Difesa, che non vuol dire stanziamenti per le Forze armate, ma stanziamenti a difesa dei nostri valori. È questo il senso del sacrificio del Milite Ignoto, almeno nella mia visione. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes.

i cento anni da quel percorso così doloroso, ma così importante per l'Italia di quel tempo, che fece quel treno, percorrendo tutto il Paese con decine,

si trattava di decidere a chi spettasse, ad esempio, la scelta della salma. Non tutte le Nazioni hanno scelto una madre; anzi, solo l'Italia ha scelto una madre. Ci furono Nazioni che scelsero un generale, altre scelsero un militare decorato al valor militare e credo che qualcuna scelse un orfano. L'Italia, che fece una commissione per decidere come dare il massimo onore e a chi spettasse quella scelta, scelse una madre, che, con lo strazio nel cuore per la perdita del suo figlio amatissimo, tremante dal dolore di fronte a quelle bare ma con determinazione scelse quella che doveva essere la bara del soldato sconosciuto, ignoto, ma che rappresentava

non ricordava solo il dolore collettivo, ma anche il dolore di ogni singola famiglia, di ogni singola persona, i cari persi, i lutti, le ferite di chi era tornato dalla guerra ma non poteva più svolgere le proprie mansioni. È stata

si trovasse davvero tutto il popolo coinvolto in un conflitto, con quella terribile guerra di trincea, con quegli assalti che poi tornavano indietro, con quelle morti continue e quei valorosissimi che si buttavano fuori dalla trincea e, pur sapendo che avevano di fronte chi stava sparando, seguivano l'ordine e andavano avanti.

dei nostri eroi in armi e farlo diventare un momento di pianto collettivo, ma anche di identità nazionale. È molto bello

memore di quelle tragedie e di quei morti. Penso sia importante anche qui, nel luogo alto della rappresentanza parlamentare, fare memoria di questo, perché fare memoria è è sempre fondamentale: non esiste un futuro se non hai radici nel passato, e la storia è qualcosa di fondamentale per capire anche dove andare.

profondo ringraziamento per il fatto che oggi, in quest'Aula, ci uniamo alla commemorazione, nella giornata delle Forze armate, del centenario della istituzione del Milite Ignoto. Credo si debba dare atto del fatto che con esso si creò uno strumento attraverso il quale consentire una sorta di elaborazione del lutto all'intero Paese; un Paese che aveva subito, nel corso della Prima guerra mondiale, la perdita di ben un milione e 240.000 giovani uomini (questo è il numero stimato delle vittime), oltre 200.000 dei quali rimasero senza nome, tali da non poter essere identificati. Quindi oltre 200.000 famiglie rimasero

c'è una storia - a volte più storie - di ragazzi partiti per il fronte. Ricordo l'ultima classe chiamata al fronte che indossò quella divisa, la divisa italiana, e portò con onore le armi: la classe del 1899. Erano ragazzini e, come è stato ricordato in quest'Aula, arrivavano dalle parti più disparate della nostra Patria ed erano perlopiù provenienti da famiglie estremamente umili. Persone che lavoravano la terra, chiamate al fronte per difendere, come si diceva allora, i sacri confini della Patria. Una parola

È smentito quello che diceva Francis Fukuyama, qualche anno fa, in un suo non dimenticato libro, «La fine della storia»: la storia non finisce; la storia, purtroppo, tragicamente continua, con le sue aberrazioni e con le sue tragedie, bisogna essere pronti anche a questi eventi. Per questo dobbiamo ricordare, con sentimento di estrema e forte gratitudine, non solamente la data del 4 novembre, la festa delle Forze armate, ma i cento anni del Milite Ignoto, che li rappresenta tutti, i caduti di quella terribile guerra civile europea. Forse vincemmo quella guerra, ma perdendo la pace, perché la Seconda guerra mondiale non fu altro che la prosecuzione, tragica, della Prima guerra mondiale Ho ricordato all'inizio che nella storia di ciascuno di noi,

era al fronte e aveva conquistato, dopo tanti mesi di prima linea, una licenza. Stava per tornare a casa, a Bolzano. Sentì che il suo reparto era attaccato: tornò su per difendere i suoi commilitoni e perse la vita. Mio nonno paterno, invece, era capitano medico nella Prima guerra mondiale. Quindi, sono cresciuto con due diverse identità, se vogliamo, ma in realtà è un'identità unica, perché quella tragedia colpì veramente tutta l'Europa in maniera estremamente forte. Oggi, il ricordo del Milite Ignoto in ogni città,

per le madri, quando arrivava il telegramma che annunciava una morte. Quindi, un sentimento che non è solo patriottico. Non c'è solo la Patria, ma, almeno in me, c'è anche la "matria".

con quel sentimento vero che appartiene a tutti coloro che si sentono debitori nei confronti di questa generazione che pagò un tributo altissimo alla libertà e alla pace.

mettere all'ordine del giorno questo punto importante del ricordo della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria. Il mio sarà un breve intervento, visto che non posso che ritrovarmi con tutto ciò che è stato detto finora dai colleghi sull'importanza di questo momento, che va sicuramente colto per ritrovarsi intorno ad un simbolo forte dell'unità di questo Paese. Sono intervenuto perché

che teniamo alle nostre differenze e particolarità, ma credo che sia importante ritrovarsi, anche da parte nostra, intorno a questi simboli forti. Intervengo soprattutto per ricordare come la Valle d'Aosta, che rappresento,

l'unico battaglione alpino decorato con la medaglia d'oro al valor militare, decorazione che fu data alla bandiera di guerra del IV Reggimento alpini semplicemente perché fu uno dei battaglioni

a vedere le lapidi in tutti i Comuni si trova un numero incredibile di giovani che hanno perso la vita in quel conflitto in quel conflitto mondiale. Anche noi, quindi, ci ritroviamo in questo momento a ricordare questo episodio, soprattutto come monito

dall'altra parte se oggi abbiamo la pace è perché tanti anni fa i nostri nonni e i nostri bisnonni si sono sacrificati fino alla morte. Credo che al termine degli interventi che hanno voluto ricordare il centenario dell'arrivo del Milite Ignoto a Roma, sia giusto, come ha fatto la Camera dei deputati, dedicare al Milite Ignoto, ma anche a tutti i caduti della Prima guerra mondiale, anzi ai caduti di tutte le guerre, senza distinzione di divisa, di

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Romeo.

Prendiamo atto, ma non siamo d'accordo sul fatto che si continui su questa strada, soprattutto con il ricorso a tale strumento, anche quando, nei vari provvedimenti, gli emendamenti sono davvero pochi (in questo caso trenta), e potrebbero essere votati in poco tempo. È vero che c'era la richiesta di un voto segreto, ma il Parlamento è questo, signori: ci sono i voti, ci sono i voti segreti, ci sono i Regolamenti, questa è la democrazia.

il Parlamento, che è composto dai rappresentanti del popolo, come se diventasse una sorta di fastidio andare in Parlamento ad affrontare le varie tematiche. Questa non la reputiamo essere una cosa giusta e corretta. In certi casi, di fronte a numerosi emendamenti e a un certo tipo di ostruzionismo, può essere anche giustificato; ma il ricorso a uno strumento del genere su tutti i provvedimenti non lo riteniamo utile. Noi ci

Guardate che l'insofferenza non è solo della Lega, che magari non è capace di nascondere certe cose, perché, forse

Presidente, mi collego al ragionamento svolto dal capogruppo della Lega Romeo, che apprezzo e condivido; naturalmente avrei piacere che ne traeste anche le conseguenze da questo assurdo ricorso al voto di fiducia. Signor Presidente, io sono uno di coloro che orgogliosamente e fieramente ha contribuito ad affossare il disegno la scorsa settimana e per questo sono stato anche pesantemente minacciato, tanto da dover presentare denuncia alla Polizia postale. Bene, oggi cosa succede? Nel momento in cui noi fieramente abbiamo bloccato quel disegno di legge, nel momento in cui noi abbiamo fieramente impedito che si arrivasse a un diritto penale dello stato d'animo interiore, come detto chiaramente dal nostro capogruppo in Commissione giustizia Balboni,

facendo entrare dalla finestra quello che è stato fatto uscire o al quale era stato impedito di entrare dalla porta. Signor Presidente, noi ci chiediamo come sia possibile

discriminatori in riferimento all'orientamento sessuale. In sostanza, una mamma che accudisce il bambino potrebbe essere ritenuta uno stereotipo di genere e potrebbe esserne

poteva prevedere una norma che non facesse arricchire qualche famiglia italiana sulla vicenda delle autostrade. Altro che riprodurre il disegno di legge Zan in un decreto trasporti! Allora, signor Presidente, chiediamo al Governo Draghi di non essere complice di queste cose; chiediamo ai partiti del centrodestra, a coloro

di dire basta a questo ricorso indiscriminato al voto di fiducia. Basta prendere in giro il Parlamento! Erano 30 emendamenti e nemmeno quelli avete voluto affrontare in Parlamento! Presidente Draghi, questa rimane comunque una Repubblica parlamentare. Non so se qualcuno ha in mente di farla diventare Presidente della Repubblica mantenendo anche il ruolo di Presidente del Consiglio, io però per ora la invito a ricordarsi che il Parlamento ha delle prerogative a cui non intendiamo abdicare, e che Fratelli d'Italia rimarrà ferma nel nel difendere il Parlamento, le sue prerogative e la libertà degli italiani contro ogni autoritarismo che non accettiamo e non accetteremo mai. senatore De Falco.

Il Governo alla 8a Commissione del Senato ha risposto tramite il proprio Sottosegretario ai trasporti che il Parlamento non può vedere e non può conoscere quell'atto. Colleghi, stiamo trasformando in legge un atto sulla base di un presupposto che non possiamo conoscere.

i lavoratori non passano all'imprenditore cessionario se questa vendita d'azienda la chiamiamo diversamente, ovvero la chiamiamo vendita di parti, vendita di compendio, vendita di parti del compendio. fingiamo che sia la vendita di parti e non di un'azienda e, quindi, evitiamo che passi anche il contratto del lavoratore dipendente dell'azienda. si mortifica totalmente il diritto del lavoratore; si annullano le relazioni sindacali. Questo è un paradigma che stanno inserendo nel nostro ordinamento attraverso una nota che traduce in legge un atto segreto. È ignobile; è una violazione della Costituzione nella formazione della legge ed è una violazione dei diritti fondamentali del lavoratore in essere. È un paradigma che si crea e che si estenderà domani al ramo di azienda *handling*, dopodomani alla manutenzione e poi, evidentemente, a tutti i rapporti di lavoro. a tutti i rapporti di lavoro. Così torneremo all'Ottocento, quando il lavoratore era solo e nudo, con le proprie esigenze, la propria famiglia e i propri bisogni, davanti ad un datore di lavoro padrone,

Purtroppo nella quotidianità spesso non si rilevano i fatti che man mano diventano sempre più critici, proprio in virtù della loro quotidianità. In realtà ci sono degli avvenimenti, che stanno accadendo in questi giorni, che lasciano veramente perplessi, come il provvedimento opposto

la funzione dei commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma, ce n'è uno in particolare, che era già stato presentato alla Camera dei deputati dai colleghi Varchi, Trancassini e Prisco,

sono differenti e l'intervento che deve essere fatto in Italia e che dovrebbe essere univoco in realtà viene differenziato in base alle aree geografiche. Non solo; un terremoto è un terremoto o dipende dall'estensione geografica del danno? È necessario che vi siano delle vittime sacrificali per ritenerlo tale e quindi richiedere un intervento immediato? [**Presidenza del vice presidente

della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'obiettivo era quello di fare una legge quadro, quindi una legge di intervento da adattare a tutto il territorio nazionale.

dal sisma. Al di là del rapporto personale, arrivo al merito della questione che è proprio politica. Il MoVimento 5 Stelle che, ad esempio, su Catania e provincia ha nominato il commissario alla ricostruzione,

Il provvedimento cui facciamo riferimento e di cui chiediamo l'estensione, oltre a prevedere la nomina dei due commissari, estende la

e quant'altro. Senza poi sottodimensionare o comunque non tener conto di quanto già riferito dal senatore Malan ieri e oggi dal senatore De Bertoldi

le due vicende hanno la medesima radice, cioè quella di negare anche l'evidenza di fronte alla ragione

e non si capisce bene dov'è andata a finire tutta questa enorme massa di danaro spesa anche dalle due gestioni commissariali.

IVA. Si potrebbe andare avanti a dismisura con i numeri per illustrare ai colleghi l'assurdità di una decisione che arriva all'epilogo di un lungo percorso a negare la possibilità di indagare da parte del Senato della Repubblica su quello che accadde nella gestione di questa emergenza. Due circostanze aggravano il tema. La prima è che tutti i grandi Paesi d'Europa hanno istituito Commissioni di inchiesta, alcune delle quali hanno già esaurito il loro lavoro e riconsegnato alle Assemblee parlamentari il frutto del loro lavoro: mi riferisco al Regno Unito, alla Spagna, alla Francia. alcune Regioni (le più grandi, ma anche alcune piccole) hanno istituito Commissioni d'inchiesta regionali sulla risposta dei servizi sanitari regionali all'emergenza Covid-19. Vi sono poi altre evidenze. In ogni legislatura (almeno nelle ultime quattro o cinque) è stata istituita una Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale,

ma viene confezionato alla stessa stregua, e viene depositato "prendere o lasciare" senza dibattito, apponendo la questione di fiducia anche su 30 emendamenti, come diceva poco fa il collega De Bertoldi. Rispetto a queste evidenze

arriva il Covid, evidentemente ad aggravare il quadro e ad accentuare la necessità di vedere che cosa accade nella materia complessiva della gestione dell'emergenza e in particolare nella risposta dei provvedimenti

Non volete essere sinceri sulla circostanza che non ci sono le carte in regola, per cui non si può andare a indagare i mille fatti oscuri di questa vicenda, a cominciare dai contratti di fornitura dei vaccini, secretati? Ne dico una, ma ne potrei dire cento. Trovate altre scuse, trovate altri argomenti. Non vi presentate davanti ai cittadini con questo argomento, perché è evidente che nessuno può comprendere che cosa sta accadendo e la distanza

dal clamore dei centri di potere. Questi familiari hanno chiesto una sola cosa, che il Parlamento indaghi sul Covid, su quello che è accaduto e su quello che sta accadendo.

quello che accadrà nei prossimi giorni, perché Fratelli d'Italia ha chiesto al Governo di venire in Aula a discutere di questa vicenda e di questa richiesta. Richiamo tutti a un senso maggiore di responsabilità e di consapevolezza del nostro ruolo di senatori della Repubblica.

signor rappresentante del Governo, il quale sicuramente è degnamente rappresentato, ma visto che un Ministro viene a mettere la fiducia, forse se ascoltasse anche quello che dice il Senato, visto che il Senato è privato di qualunque possibilità di intervenire, non sarebbe male.

In quella lettera si citava il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, che ha invitato il legislatore a evitare la commistione e la sovrapposizione nello stesso atto normativo di oggetti e finalità eterogenei.

per materia; nei casi in cui l'omogeneità sia perseguita attraverso l'indicazione di uno scopo, deve evitarsi che la finalità risulti estremamente ampia. Il Capo dello Stato prosegue osservando che: nella procedura di conversione l'attività emendativa dovrà essere limitata dalla materia, ovvero dalla finalità originariamente oggetto del provvedimento, come definite dal Governo. Ricorda infine, insieme a molte altre osservazioni che non possiamo certamente leggere tutte qui, con la sentenza n. 32 del 2014, la Corte costituzionale, dichiarando illegittime alcune norme introdotte in sede di conversione di un decreto-legge, ha sottolineato che la legge di conversione

e che dalla sua connotazione derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge; la legge di conversione non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore. Questo il messaggio del Presidente della Repubblica tutta la maggioranza e naturalmente anche noi rispettiamo profondamente, ma la maggioranza di solito è particolarmente accorata nel professare l'assoluta adesione alle parole del Presidente della Repubblica.

delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale; ebbene, in questo disegno di legge sulla sicurezza delle infrastrutture viene inserita una norma ideologica volta a limitare la libertà di espressione, con il pretesto che tale limitazione viene esercitata sulle strade e sui veicoli. Si tratta di una misura assolutamente inaccettabile, introdotta a tradimento e di soppiatto, tanto è vero che gli stessi proponenti dell'emendamento presentato alla Camera dei deputati (le Presidenti delle Commissioni ambiente e trasporti), entrambe del Partito Democratico, non hanno neppure illustrato il provvedimento, salvo cambiarlo per peggiorarlo nel corso del suo esame. del suo esame. Questa incredibile limitazione alla libertà di espressione è pericolosissima perché lasciata, per un verso, all'interpretazione, e per un altro, alla censura preventiva che faranno tutti i concessionari di pubblicità. Questi ultimi, per evitare problemi, saranno ancora più severi di quanto lo sarebbe un giudice o qualunque autorità deputata a pronunciarsi su cos'è una pubblicità sessista o su cosa, in un contenuto pubblicitario, potrebbe offendere qualcuno nel suo credo religioso (ad esempio, esprimendo esprimendo convinzioni di un altro credo religioso), oppure su cosa può offendere qualcuno rispetto all'identità di genere. Un concetto, quest'ultimo, ampiamente criticato quando inserito nel disegno di legge Zan, anche da parte di chi sosteneva il resto di quel provvedimento (che noi non

per un ulteriore passaggio alla Camera per eliminare questo obbrobrio, questo abuso, questa beffa alla volontà del Senato, e in particolare dei 154 senatori che, una settimana fa, hanno votato per non proseguire l'esame del disegno di legge Zan.

in questo senso: Partito Democratico, Italia Viva, MoVimento 5 Stelle, Per le Autonomie, non lo sappiamo, ma almeno 20 ci sono stati. *(Applausi)*. È dunque una beffa anche per loro, uno sfregio a loro e al popolo che essi, come tutti noi, rappresentano.

farli passare a viso aperto e non chiudere la bocca ancora una volta a tutti i senatori, in particolare a quelli della maggioranza. Come Gruppo Fratelli d'Italia, infatti, noi parliamo lo stesso, esercitando un'operazione patriottica e responsabile

ripeto, è uno sfregio al ruolo del Parlamento e alla Costituzione che affida al Parlamento il compito di fare leggi e non di fare giusto da passacarte al Governo che adotta i decreti-legge e fa inserire poi da suoi parlamentari delle norme che nulla c'entrano, ponendo infine la questione di fiducia, sia alla Camera che al Senato, per cui in pratica tutto è stato deciso dalla cinquantina di parlamentari della Commissione della Camera e per il resto non è stato più possibile fare assolutamente nulla. Come hanno detto i colleghi intervenuti - la senatrice Drago e i senatori Zaffini e De Bertoldi - c'è qui un complesso di cose che vanno tutte nella stessa direzione: schiacciare e comprimere i diritti del Parlamento

sono andato a vedere quando è stato approvato l'articolo 2112 del codice civile, che è molto moderno: si parla di trasferimento di azienda, per cui ero convinto che fosse recente. È stato approvato nel 1942: in pratica è rimasto invariato, salvo una piccola modifica di carattere tecnico nel 1990. Oggi il Governo lo cancella, danneggiando i diritti dei lavoratori di Alitalia, e un domani chissà di quante altre aziende, con un provvedimento d'urgenza su cui il Parlamento non può discutere. Seguono i sindacalisti con il foglio di via, che non possono entrare a Roma, pur avendo intenzioni del tutto pacifiche; seguono le manifestazioni vietate, spostate e deviate lontanissimo

portare all'attenzione anche della cittadinanza e degli italiani la gravissima modifica costituzionale di fatto che negli ultimi decenni si è venuta sempre più a definire e a stabilizzare. Ciò è stato perché la nostra Costituzione ha delle regole molto precise

messa in atto una modifica costituzionale di fatto. Ieri, in una interessante conferenza stampa promossa dal senatore De Falco, l'avvocato Anna Falcone Anna Falcone ha detto in maniera molto semplice - a volte le frasi semplici arrivano più direttamente - che il Parlamento dovrebbe controllare il Governo: ciò è alla base della nostra Costituzione, è l'architettura; più volte ha parlato di «architettura», perché è una costruzione che sta in equilibrio, che si basa sulla divisione dei poteri per stabilire la democrazia; tutte parole di cui noi facciamo amplissimo uso e abuso, realtà il Parlamento non controlla più niente. Le funzioni delle Camere, che dovrebbero sostenere e dare la fiducia, non sono più da tempo quelle del controllore

e, quindi, va controllato da tutti gli italiani. Ebbene, questo non avviene più. Per qualunque cosa - e vi posso dire a ragione vale anche per i disegni di legge di iniziativa parlamentare - si cerca sempre e comunque il controllo governativo. Per tutti i pareri che le Commissioni esprimono sugli atti del Governo - adesso ci siamo ridotti a dare dei pareri - ci troviamo a chiedere al Governo se l'espressione che abbiamo usato nel nostro parere sia consona;

nella Commissione competente per quarantotto ore, è l'articolo 7 che - è stato detto, ma lo voglio dire anch'io riesce ad aggirare l'articolo 2112 del codice civile sulla tutela dei lavoratori e delle relazioni sindacali. Si crea un precedente pericolosissimo, perché liquida uno dei comparti più importanti del nostro Paese - ad oggi i lavoratori Ilva sono circa 8.000 - con l'articolo di un decreto-legge su cui viene posta la fiducia. Si è già pensato più volte di superare il fatto che nella cessione di azienda chi acquisisce deve prendersi anche i contratti dei lavoratori. Ma si è trovato

il tentativo di Renzi, fermato dalla Cassazione, oggi passano con un voto di fiducia. Ciò è enormemente grave ed è anche un'aberrazione che avvantaggia altri Stati

Signor Presidente, ancora una volta un ramo del Parlamento si ritrova a dover parlare del lavoro svolto dai colleghi dell'altra Camera senza possibilità alcuna di di intervenire sul provvedimento. A me tutto questo continua - lo dico sempre e lo ribadisco - a sembrare assurdo. Se è vero che da qui alla fine dell'anno c'è tanto da fare, non è possibile licenziare provvedimenti di tale importanza in maniera così frettolosa. Anche oggi, l'unica cosa che si può fare è è salutare il lavoro dei colleghi della Camera, che hanno apportato migliorie significative a un decreto-legge complesso e ambizioso: complesso perché prevede interventi dal settore autostradale a quello idrico, da quello ferroviario a quello marittimo; ambizioso perché - da un lato - punta a semplificare e - dall'altro - guarda al tema della sicurezza e alla necessità di incentivare la mobilità sostenibile. In questa cornice sono tante le novità degne di nota, dagli interventi sul codice della strada, con l'inasprimento delle sanzioni, a quelli sui parcheggi, con un occhio di riguardo per quelle categorie per cui l'uso dell'automobile, più che una scelta, è una necessità, come le donne in gravidanza, le famiglie con bambini piccoli e i disabili; dall'attenzione per i pedoni ai finanziamenti ai Comuni per la messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana; dalle norme sulla messa in sicurezza della fauna selvatica e degli animali randagi a quelle per il decoro urbano, con la rimozione dei rifiuti abbandonati; dalle norme sull'autotrasporto alla prima vera disciplina sull'uso dei monopattini, che stanno cambiando la mobilità, soprattutto nei grandi centri urbani, ma che richiedevano una normativa sulla velocità, contro i parcheggi selvaggi, sull'uso del casco per i minori e, in prospettiva, sull'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile. Ma ancora più importante è l'impulso che viene dato allo sblocco dei cantieri, per rimettere al centro quelle opere su cui l'Italia ha perso troppo tempo e che, invece, sono un elemento essenziale per la ripartenza del Paese.

Eppure, basta scorrere l'elenco per rendersi conto che, accanto a opere strategiche, come la Torino-Lione, ci sono numerosi interventi che puntano a ripristinare condizioni di viabilità e sicurezza degne di questo nome, soprattutto nelle aree interne. Sempre su questo fronte, come Gruppo per le Autonomie salutiamo favorevolmente due novità. La prima è quella contenuta nell'articolo 16, sulla disciplina relativa alla realizzazione delle opere collegate alle Olimpiadi di Cortina del 2026, prevedendo, tra le altre cose, la possibilità, per le opere caratterizzate da elevata complessità progettuale o procedurale, il ricorso a quanto previsto dall'articolo 44 dell'ultimo decreto-legge semplificazioni. La seconda novità riguarda l'A22, con l'emendamento approvato alla Camera, che rappresenta un'importante tappa rispetto all'obiettivo più volte auspicato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'affidamento e la gestione di un'infrastruttura di straordinarie importanza

Pensiamo solo al fatto che la città di Bolzano è tagliata in mezzo da questa autostrada o al fatto che da Bolzano fino al confine quasi tutti i chilometri sono su viadotti, ponendo questioni di delicatezza ambientale e di sicurezza. La A22 La A22 fino ad oggi è stata gestita e governata in maniera esemplare dalla A22 SpA, una società all'86 per cento pubblica, di proprietà degli enti territoriali. e impensabile che la guida e la gestione di una tratta autostradale essenziale, delicatissima per tutto il territorio italiano - parliamo della tratta più importante, da Nord

non ha alcun rapporto. Sarebbe inspiegabile e non sarebbe responsabile. Pertanto, noi speriamo tanto che, con questo provvedimento, si riesca ad affidare finalmente in via definitiva la A22 alla società Autostrada del Brennero. Vi sono, poi, altre norme importanti, come quelle su ANAS e sulla nuova compagnia di bandiera. Vi sono tutte le importanti novità procedurali connesse alla progettazione delle opere, ai commissari, al ruolo di Cassa depositi e prestiti e di Mediocredito centrale per l'assistenza e il supporto operativo alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione del PNRR. Tutto questo, signor Presidente, serve a ribadire l'importanza del provvedimento, le buone norme che vengono introdotte, ma anche il fatto che il Senato non meritava di ridursi a una funzione di passacarte. Fatte tutte queste considerazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento. il provvedimento che ci apprestiamo a votare è, sostanzialmente, un decreto *omnibus* sul tema delle infrastrutture, della mobilità e della circolazione stradale. Prima di entrare nel merito del problema del provvedimento, mi vorrei soffermare su una premessa metodologica e di lavoro. Si tratta di un decreto nato dall'esigenza di raccogliere le tante sollecitazioni provenienti dai più svariati ambienti e che, proprio per la modalità con cui è stato pensato e poi venuto alla luce, aveva fin da subito un limite, ossia quello di non avere un *fil rouge* definito. Il grande lavoro fatto anche dai colleghi della Camera è andato proprio in questo senso. Devo dire che è stato un lavoro che si è concluso portando importanti frutti. frutti. Quello che ci troviamo oggi ad approvare e a convertire in legge è un decreto che, sebbene nasca dall'unione di molti interventi e svariate misure, il cui nesso non è da subito risultato immediato, ha trovato una sua direzione e una sua specificità. Nel quadro del corposo lavoro fatto, gli sforzi sono stati congiunti, da parte di maggioranza e di opposizione. Questo *modus operandi* è un importante segnale per il lavoro cui noi tutti siamo chiamati e in cui saremo sempre più impegnati nei prossimi mesi. Devo, però, anche operare una considerazione di rammarico su un aspetto. Pur comprendendo lo sforzo profuso dai colleghi della Camera e le tempistiche fortemente contingentate, dettate dalla conversione di un decreto-legge, auspico che l'esame dei futuri provvedimenti possa essere portato avanti in maniera approfondita da entrambi i rami del Parlamento. Venendo al merito del provvedimento e volendo schematizzare il contenuto complessivo del decreto, i temi centrali su cui si innestano le misure che ci accingiamo a votare potrebbero essere due: sicurezza e semplificazione. Penso - ad esempio - all'introduzione nel codice della strada degli stalli rosa, per il parcheggio delle donne in gravidanza e i genitori con i figli fino a due anni di età, e il rafforzamento delle sanzioni per chi occupa i parcheggi riservati senza essere autorizzato. alla possibilità per le Regioni di utilizzare una quota delle risorse erogate per i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale anche per potenziare i controlli. Per il miglioramento della rete ferroviaria sono state confermate le norme per accelerare l'attuazione del Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico, cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza assegna importanti investimenti. Il decreto rafforza, poi, il ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, per migliorare efficacia ed efficienza del sistema dei controlli. Confermata anche la disposizione volta ad agevolare gli investimenti per ridurre i divari infrastrutturali su tutto il territorio. Da questo breve cenno al contenuto del provvedimento, si può facilmente intuire che si tratta di un decreto che reca in sé misure di semplificazione che contribuiscono anche al buon esito del PNRR, sul quale il Governo sta lavorando con impegno e fruttuosamente. Mi piace anche dire che queste misure si inseriscono nel solco delle richieste che da tempo Italia Viva avanza. E faccio riferimento al piano *shock* per le infrastrutture e alla contestuale necessità di sbloccare tutte le opere. Occorre comprendere che la ripartenza di questo Paese passa attraverso la sua infrastrutturazione fisica e digitale. Dunque, il decreto-legge che ci apprestiamo ad approvare va nella giusta direzione, ossia in una direzione competitiva, nell'ottica della ripartenza economica e lavorativa del Paese, ma anche in quella del migliore utilizzo del PNRR. Le infrastrutture ed i trasporti rappresentano uno dei terreni su cui, come Paese, siamo chiamati ad intervenire con maggiori finanziamenti e più incisive migliorie. Sotto il primo profilo, il mio auspicio e quello del Gruppo che rappresento è che le coperture economiche, che son risultate per certi versi deficitarie in questo decreto-legge, possano invece trovare una sede nella legge di bilancio che nelle prossime settimane saremo chiamati ad esaminare. Sotto il secondo profilo, ossia quello del miglioramento, credo che si debba e si possa fare ancora molto. Penso - ad esempio - al delicato settore della sicurezza stradale: nonostante la forte riduzione del traffico automobilistico, derivata dal periodo emergenziale, non si è avvertita una parallela riduzione degli incidenti stradali. Allo stesso modo, la sicurezza dev'essere preservata anche per uno strumento che, specialmente durante la pandemia, è risultato molto utile e mi riferisco ai monopattini. La comodità di un simile strumento però deve necessariamente passare in secondo piano rispetto alla sicurezza: lo dice espressamente anche lo stesso testo del decreto, dopo le modificazioni che sono state apportate. Leggo testualmente: «La sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché la tutela dell'ambiente nella circolazione stradale rientrano tra le finalità primaria di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato». È quello che abbiamo cercato di fare nel nostro piccolo e attraverso l'operato prezioso dei colleghi della Camera. Quella dei monopattini elettrici rappresenta sicuramente un'innovazione anche ambientale per le nostra città e, quindi, deve essere salvaguardata e preservata. Naturalmente, però, vi deve corrispondere una capacità di monitoraggio rispetto alla sicurezza, che deve invece essere rafforzata. contribuire alla transizione ecologica del Paese anche attraverso questi strumenti, ma è necessario farlo in maniera intelligente e soprattutto rispettosa delle regole. Un altro settore su cui occorre intervenire in maniera ancora più decisa riguarda quelle che potrebbero essere definite come norme di civiltà. Penso - ad esempio - al permesso rosa, che riguarda le donne in gravidanza e i primi due anni della maternità. Nello stesso solco, anche se in maniera diversa, si inserisce il divieto sulle strade e sui veicoli di qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o discriminatori. Sotto altro specifico profilo, vorrei sottolineare l'importante lavoro fatto dalle colleghe di Italia Viva della Camera a tutela delle persone con disabilità. Ad un inasprimento delle sanzioni per l'occupazione dei parcheggi riservati da parte di soggetti non autorizzati, si affianca anche la possibilità per le persone con disabilità di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu qualora risultino occupati i parcheggi a loro riservati. Credo poi che ci siano altri temi prioritari da mettere in agenda quanto prima perché necessitano di riforme organiche: il trasporto pubblico locale, che deve essere completamente rivisto nella sua disciplina e che deve guardare con maggiore attenzione agli utenti; maggiori e più incisivi interventi di semplificazione anche nell'ottica della attuazione concreta del PNRR; il rafforzamento delle strutture commissariali, che sono state per il momento solo individuate. Questi sono solo alcuni aspetti che il decreto che oggi ci apprestiamo a convertire non può prendere in considerazione, anche perché necessitano di una visione di più ampio respiro. Credo però

Sono quindi particolarmente contento che questo decreto-legge rappresenti un primo tassello di un *puzzle* molto più ampio, che noi tutti siamo chiamati a comporre, perché riguarda obiettivi di lungo periodo che rappresentano una grande scommessa sulle infrastrutture, sulla ripresa, sulla ripartenza economica e e sul lavoro. Per tutte queste ragioni, il voto di Italia Viva-PSI non può che essere convintamente a favore. *(Applausi)*.

di questo ennesimo decreto-legge *omnibus* - stavolta, tra l'altro, tra i più corposi e variegati - che tratta una *summa* che va dalle autostrade alle ferrovie, dal trasporto marittimo ai monopattini e all'extrabonus per i veicoli elettrici. Addirittura il parco della giustizia di Bari - non che non sia importante - viene inserito in questo enciclopedico processo. Ci sono poi le nuove identità digitali, le misure per i Comuni l'emergenza epidemiologica, la Protezione civile per le isole minori, gli asili nido, il sistema portuale dello Stretto di Messina - come ricordava la nostra senatrice Drago - il ponte Morandi. Meritavano quantomeno la possibilità di essere approfondite tutte queste grandi questioni, che interessano la vita della nostra Nazione. Tutto ciò, invece, ci dà la possibilità di una riflessione, l'ennesima, non più rinviabile, sull'impalcatura dello Stato, sul senso stesso delle Commissioni e sul ruolo dei commissari. Poteva essere l'occasione, per il tanto celebrato Governo dei migliori, di di affrontare la questione. E, invece, il Governo dei migliori, pur avendo la più grande maggioranza parlamentare che la storia ricordi, si comporta perfettamente in continuità con i Governi passati

proposto da Fratelli d'Italia con il voto segreto. Ciò vi consente però di concorrere a

siete forti con i deboli e deboli con i forti; duri, durissimi con i lavoratori dell'Alitalia, sui quali si scaricano senza alcuna pietà gli errori del passato, come nella peggiore tradizione neoliberista; morbidi, morbidissimi con i padroni, con la famiglia Benetton, al di là dei proclami. Sapete cosa sta accadendo al riguardo? Si sta strapagando la quota che i Benetton hanno in Autostrade per l'Italia, quando ci si potrebbe avvalere del diritto di recesso che è previsto dalla convenzione. Non è una cosa da poco: si spenderebbero 13 miliardi anziché 21. Gli 8 miliardi in più li pagheranno come al solito gli automobilisti italiani e il sistema Italia. Governo è forte con i lavoratori e debole con i padroni, come è successo con ITA e nei confronti dell'Europa, che ancora una volta nega all'Italia quello che ha fatto per la Francia e per la Germania. A differenza di Francia e Germania, noi abbiamo dato spazio e linfa vitale alle *low cost*; Francia e Germania le hanno tenute sapientemente lontane dagli aeroporti importanti. Quindi, ITA partirà con risorse per reggere un paio di inverni in perdita; poi arrivederci al prossimo Governo. Povera Italia. Altro che Governo dei migliori!

conoscenza dai telegiornali delle tragedie avvenute. Abbiamo chiesto con i nostri emendamenti un'adeguata regolamentazione del codice della strada o una copertura assicurativa necessaria anche per i privati.

è poi una questione alla quale Fratelli d'Italia tiene molto. Mi riferisco alle patenti. Al di là delle grandi questioni, in Italia mancano circa 5.000 autisti, numero che arriverà a 17.000 nel prossimo biennio. Il nostro territorio pullula di vettori stranieri; le nostre strade sono percorse da aziende di autisti che agiscono - secondo noi - in un clima di concorrenza sleale

l'interessante emendamento per gli amanti del *gossip* inserito tra le disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti.

Evito di leggere il contenuto dell'articolo perché, dietro una patina così politicamente corretta, sappiamo bene che cosa si nasconde.

Signor Presidente, rivolgo un ringraziamento al relatore senatore Astorre, che, seppure in condizioni delle quali parlerò adesso, in due giorni ha svolto un ottimo lavoro. Le condizioni sono quelle di un monocameralismo di fatto. L'hanno detto già quasi tutti i colleghi intervenuti. Non è una novità di questa legislatura e di questo di questo Governo, ma via via che passa il tempo esso diventa sempre più vigente. Invece del bicameralismo perfetto, mi pare che siamo al monocameralismo imperfetto. la riforma costituzionale del 2016 poteva essere un modo di superare e migliorare una situazione di siffatto tipo. C'è una piccola consolazione, ma solo per i deputati. Alcuni degli articoli che il Governo aveva inserito nel decreto iniziale corrispondono a richieste approvate ai primi di agosto di quest'anno attraverso un ordine del giorno fatto alla Camera e che poi è diventato traccia di lavoro per il Governo. Si tratta di un decreto *omnibus*. Ha tantissimi aspetti ed elencarli tutti sarebbe esercizio vano. Mi soffermerò solo su alcune delle cose che ritengo maggiormente positive. Proprio in quanto decreto *omnibus* ci sarebbe piaciuto poterci lavorare anche al Senato.

disposizione legislativa su una serie di norme, che correggono e migliorano il codice, sia stata una scelta importante. Allo stesso modo voglio sottolineare l'utile lavoro fatto in materia di autorità portuali, con una serie di interventi, tra cui mi piace citare una questione apparentemente minore, ma che tale non è, che è quella del cosiddetto recupero dei relitti di navi: ce ne sono infatti tanti nei porti italiani. Molto positivo è il fondo per la progettazione nelle zone svantaggiate, ovvero quelle interessate dall'Agenzia per la coesione territoriale. Solo dotando per tempo le amministrazioni di progetti validi, dunque di una sorta di parco progetti, potranno essere sfruttati appieno i diversi finanziamenti compresi nel PNRR e non solo: vedremo che nella legge di bilancio, che tra poco sarà all'esame di questo ramo del Parlamento, c'è un'importante previsione di ulteriori fondi da investire nelle infrastrutture. Sono importanti anche le disposizioni in materia di Piano nazionale di interventi nel settore idrico, a cui il PNRR dedica finanziamenti molto rilevanti, tanto per il settore della grande adduzione, della distribuzione, delle reti e dei sistemi irrigui, quanto per quello delle fognature e della depurazione. Vi sono misure in materia di formazione e attuazione del piano di monitoraggio e, soprattutto, poteri sostitutivi nel caso di inerzia di alcune amministrazioni.

il settore dei trasporti e della logistica, pur essendo quello più colpito, è stato anche quello che ha reagito meglio, non abbandonando mai gli italiani che si potevano muovere

tanto una commissione insediata dallo scorso Governo: il testo c'è e bisognerebbe accelerare per analizzarlo, perché si tratta di un tema molto importante. Ho qualche dubbio sull'Anas, che viene sdoppiata, creando una nuova società che si occupa di tutte le strade a pedaggio, che esce dal perimetro di Ferrovie dello Stato e va sotto la

che non è a pedaggio. Non vorrei che questa parte diventi una sorta di *bad company* e l'altra diventi la *newco* in materia di strade. In ogni caso, c'è un'inversione netta rispetto alla visione della scorsa legislatura, quando invece si ritenne importante immettere ANAS in Ferrovie dello Stato con un disegno organico obiettivamente diverso da quello che è stato poi realizzato in questo tempo. È una scommessa, e vedremo come va. Sul punto mantengo qualche perplessità, così come le mantengo sui provvedimenti in materia di trasporto aereo. Tutta la vicenda che riguarda Ita e Alitalia ha ancora molte ombre, almeno per quanto mi riguarda, e devo dire che le audizioni del *management* nelle Commissioni competenti non hanno per nulla

spero che sarà il Senato a poter avere la prima parola in modo da lavorarci tutti insieme, nel modo migliore possibile. Nel frattempo accontentiamoci di ciò che è stato fatto, che non è poco, è ed è anche il motivo per cui il Gruppo Partito Democratico esprimerà

Trovo positivo e significativo che si siano fatte alcune scelte. Penso - ad esempio - al piano per la sicurezza nel settore idrico, grande tema che esprime una situazione sempre più drammatica nel nostro Paese, anche in relazione al cambio climatico, che richiede una

valorizzare la risorsa acqua e di gestire al meglio le situazioni di criticità su interventi di grande significato per l'assetto idrogeologico del nostro Paese. I dati anche dell'ultimo piano, pubblicati recentemente, ci dicono però che, rispetto alle potenzialità di spesa, siamo non oltre il 25 per cento. Bisognerà pure che, a partire dal Governo, si prenda atto che qualcosa non va nel modo di gestire

Da questo punto di vista un segnale positivo, grazie al lavoro svolto alla Camera, arriva dal Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, che recupera anche - come qualche collega ha sottolineato - la situazione del Centro Italia, che appare problematica anche in relazione alle scelte di priorità che il Governo ha fatto e deve fare. Consentitemi di aprire una parentesi ed esprimere sinceramente in quest'Aula una preoccupazione: è un segnale importante e positivo, ma non stiamo prendendo atto con la coerenza necessaria del fatto che la struttura pubblica, la pubblica amministrazione nel nostro Paese, mostra una carenza drammatica nella capacità di progettazione, di gestione delle gare e delle opere pubbliche.

dei fondi, ma i nodi verranno al pettine e rincorrere questa carenza drammatica,

a sostenere la ripresa del nostro Paese. Allo stesso modo trovo importante, ma forse ancora timida, la regolazione del tema dei monopattini, che è una grande questione relativa alla sicurezza. Non è stato approvato l'obbligo del casco, ma in questa sede

quale vogliamo dedicare due sollecitazioni al Governo. Mi riferisco all'articolo 7, in relazione al tema di Alitalia.

che possono rappresentare un problema molto serio e significativo per il futuro, nella gestione di un tema relativo alle relazioni industriali, che richiederebbero in verità un passo in avanti di qualificazione per gestire questa nuova fase (la transizione ecologica, la rivoluzione tecnologica). In verità in questo caso si sta facendo un grave passo indietro.

molti Gruppi già hanno sollevato: si devono programmare i lavori del Governo e rispettare l'autonomia del Parlamento.

così ristretti e che non ci sia nemmeno il modo di valutare gli emendamenti, anche perché, fatta la lettura in una Camera, la seconda lettura non esiste più. Poi magari ci troveremo a discutere del bilancio e ci si dirà che dobbiamo fare le tre letture. In verità, non faremo le tre letture, ma i tempi e i modi per valutare il bilancio saranno comunque ristretti.

Presidente, colleghi, innanzitutto guardiamo al positivo e ai molti contenuti di questo decreto-legge che avranno buoni effetti sull'economia del nostro Paese. È solo per questo che Forza Italia voterà favorevolmente e sosterrà questo provvedimento. Ci sono contenuti positivi e anche ieri la collega Fiammetta Modena citava quelli relativi alla sua Regione, l'Umbria, ma lo stesso vale per molte altre Regioni che avranno vantaggi infrastrutturali. Con tutta la nostra buona volontà, colleghi, non possiamo però non essere critici per la gestione di questo provvedimento, per l'*iter* che ha seguito. Come diceva anche il collega che mi ha preceduto, ma l'hanno detto in molti, è evidente che questa ennesima manifestazione dell'attuazione di un monocameralismo alternato di fatto deve cessare;

all'ultimo momento, nella seconda lettura invece che nella prima, i temi che sono diventati urgenti e sono inseribili e il terzo passaggio si può risolvere con breve tempo, con una fiducia, come purtroppo accade anche oggi, ma questo renderebbe più dignitoso il nostro lavoro.

a meno di quarantotto ore da quando è iniziato il nostro lavoro in Commissione. Non so se è un record, forse no, ma vi assicuro che per un decreto come questo è davvero difficile da giustificare. A ciò si aggiunge il fatto, a cui altri colleghi hanno già accennato, che questo provvedimento si può definire a tutti gli effetti una via di mezzo tra un *omnibus* e un mille proroghe. C'è davvero C'è davvero un po' di tutto e questo - perdonatemi se lo dico - aggrava la situazione. Ci sono modifiche al codice della strada, è vero, molto positive in alcuni casi, che prevedono parcheggi dedicati a categorie svantaggiate. la nuova disciplina per la circolazione di monopattini, insieme a cose ben più serie come le nuove norme in materia di infrastrutture autostradali e idriche, queste ultime in particolar modo urgenti. È in È in particolar modo urgente e utile inoltre, l'introduzione della finanza di progetto. Trattiamo la delicata transizione Alitalia-ITA e non mancano i rimborsi dei componenti della commissione nazionale per il dibattito pubblico della cui esistenza vengo a sapere tramite questo provvedimento. Perdonatemi, forse sarò male informato ma non so, colleghi, quanti di voi sanno che esiste una commissione nazionale per il dibattito pubblico; prima o poi ci diranno anche di cosa si occupa perché è effettivamente particolarmente strano. Nel testo troviamo anche - ma ci sta - l'incremento di talune indennità e fondi per alcune componenti della retribuzione del personale non dirigenziale e dirigenziale del MIMS e altre questioni che dovevamo e potevamo affrontare, ma che non sono state trattate,

una sanzionabilità senza definire la sanzione, e questo è pericoloso perché oggi decidiamo che un dato comportamento è sanzionabile, ma non decidiamo come. Questo *vulnus* è pericoloso, perché tutti saremmo d'accordo a sanzionare in un certo modo, ma molti di noi - forse tutti - non sarebbero d'accordo a sanzionare con un'altra gravità. si sappia, nella confusione di questo comma 4*-bis* che va modificato, che servirà un intervento, e anche veloce, perché rischiamo di dare ai sindaci di un Comune di 500 abitanti come di un Comune di un milione di abitanti

Il Ministro degli affari esteri, se ha voluto questa competenza, se ne deve occupare, deve metterci mano *(Applausi)*, perché la trasparenza non può essere evocata

Abbiamo presentato un ordine del giorno - ringrazio il Governo per averlo accolto - nel quale specifichiamo che le *mid cap* devono essere - come previsto dalla Banca europea per gli investimenti per tutte le Nazioni

una grossa fetta di internazionalizzazione per le nostre aziende che, invece, hanno bisogno di risorse e di aiuti. Allo stesso modo, non ci possono essere determine del comitato di gestione assunto dopo l'apertura dei bandi, con i relativi elementi informativi, - bisogna essere chiari - non basta avere il requisito di imprese esportatrici, ma serve che ci sia una presenza all'estero, altrimenti (stiamo parlando di 800 milioni più 400 milioni) queste risorse non verranno utilizzate adeguatamente. Questo non possiamo permettercelo. Dopodiché, dobbiamo affrontare anche ciò che non c'è

fondi (qualche milione) per aumentare la capacità di accosto per il traghettamento nello Stretto di Messina. È una sciocchezza: bisogna fare il ponte; bisogna fare questo benedetto ponte! *(Applausi)*. a giustificare il fatto che non si affronti il tema perché divisivo. Colleghi, oggi questo tema è divisivo innanzitutto e soprattutto per i nostri cittadini del Sud,

facendo in modo che tutto concorra a non utilizzarlo. Infatti, o si mette a disposizione dei cittadini una pianificazione, con le condizioni affinché venga utilizzato, altrimenti con più coraggio si dica che il superbonus non c'è.

Come ho già detto, Forza Italia non farà mancare un sostegno responsabile a questo decreto, ma non può essere un sostegno acritico, così come non possiamo esimerci dal chiedere un di più al Governo - ci aspettiamo davvero di più perché lo dobbiamo al lavoro dei tanti italiani che in questa fase non si stanno sottraendo a un impegno appassionato per ricostruire il Paese e non possiamo mancare noi.

il provvedimento in esame è molto articolato, contenendo disposizioni complesse in materia di sicurezza, infrastrutture, trasporti e circolazione stradale. Molte delle modifiche al codice della strada previste sono in linea con quanto la Lega propone da tempo, come, ad esempio, la possibilità di effettuare presso officine esterne autorizzate le revisioni periodiche dei veicoli pesanti, l'introduzione di aree dedicate alle donne in gravidanza e alle famiglie, incentivi ai Comuni per riservare la sosta gratuita sulle strisce blu alle persone con disabilità e disposizioni in materia di circolazione di prova, che prevedano che i veicoli non immatricolati e quelli muniti di carta di circolazione possano circolare con l'autorizzazione di prova per motivi connessi a prove tecniche, sperimentali, costruttive o dimostrazioni e trasferimenti per ragioni di vendita o allestimento. Da fiero rappresentante delle aree interne e montane più disagiate dell'Appennino modenese conosco bene quali sono le criticità viarie e la carenza di infrastrutture in cui si trova, ad esempio, il distretto ceramico di Sassuolo e tutta l'area dell'indotto economico circostante come Lega conosciamo bene l'importanza degli assi di penetrazione che dovrebbero collegare rapidamente i centri produttivi con le aree più periferiche, quasi sempre sprovviste di adeguati trasporti e telecomunicazioni. Tutti i giorni tocchiamo con mano l'isolamento e il conseguente spopolamento di piccole comunità di montagna che, una volta desertificate, saranno popolate soltanto da lupi e cinghiali. Penso con affetto, nel mio collegio, ad alcune piccole comunità, Gusciola, Piandelagotti e Sant'Anna Pelago che, sebbene siano delle piccole eccellenze culturali, agricole, imprenditoriali e turistiche, sono penalizzate dall'immenso divario digitale e viario rispetto ad altre realtà. Nonostante tutto ciò, queste comunità lottano disperatamente per sopravvivere. In modo particolare, dovremmo pensare a questi cittadini e contribuenti quando ci apprestiamo a votare provvedimenti inerenti ad infrastrutture e mobilità sostenibili. Pensiamo al caso dell'Agenzia per la mobilità di Modena, che dovrebbe prendersi cura dei trasporti scolastici per le aree interne della Provincia di Modena, dove i ragazzi di alcune frazioni di alta montagna devono prendere un mezzo pubblico alle 6 del mattino per rientrare alle 16, perché non ci sono i fondi. L'Agenzia per la mobilità di Modena - abbiamo qui le risposte - dice che non si può fare nulla; non c'è nulla da fare e questi ragazzi si dovranno arrangiare almeno fino al 2022. Ebbene, da noi le gelate sono già dietro l'angolo e la neve sta arrivando, ma questo vale per tutte le aree interne di montagna di questa penisola. Dobbiamo immaginare che questi ragazzi, che hanno un diritto allo studio e quindi alla mobilità, debbono attendere al freddo e al gelo quello che non arriva o forse arriverà. Desidero comunque ricordare che, grazie a un emendamento targato Lega, anche le macchine agricole verranno classificate di interesse storico o collezionistico, purché la data di costruzione sia precedente di almeno quarant'anni a quella della richiesta di riconoscimento. Può sembrare poca cosa, ma auspico che questo sia solo l'inizio di un nuovo approccio costruttivo della politica a favore del motorismo storico, un mondo che crea un indotto di oltre due miliardi di euro e che, se tutelato e incentivato come la Lega da tempo auspica, potrà generare ulteriore ricchezza e e bellezza. Ma la politica deve anche vigilare su quanto ancora, seppure votato ed approvato da questo Parlamento, giace sulle scrivanie ministeriali: mi riferisco ad esempio ai decreti attuativi sulle targhe storiche, che da troppi mesi ancora non vedono la luce. Ogni giorno che passa non è solo un giorno mancato per questo provvedimento, ma è soprattutto un giorno di mancato introito per le casse dell'erario: ricordiamocelo bene.

Mi permetto una breve sintesi di questi undici ordini del giorno, già in parte citati anche ieri dai miei colleghi, anche se sono stati in parte riformulati o trasformati in raccomandazione dal Governo; sono tutte proposte pratiche e realizzabili in tempi rapidi.

(problema sempre sotto gli occhi di tutti i cittadini che usano un'automobile o un altro veicolo). Mi riferisco anche all'esenzione dall'obbligo di revisione per i veicoli ultratrentennali o iscritti ai registri storici che si desidera esportare, molti dei quali rischiano di essere venduti all'estero senza la dovuta radiazione della targa, con conseguente danno erariale per lo Stato. Possibile che nessuno ci abbia mai pensato? Strano. Ma noi del territorio, come Lega, recepiamo anche queste indicazioni e le portiamo in Parlamento. Mi riferisco inoltre all'esenzione dell'obbligo di revisione per i veicoli con revisione scaduta, i cui proprietari hanno la possibilità, senza incorrere in sanzioni, di recarsi tramite apposita autocertificazione presso il centro di revisione a loro più vicino; non è che una cosa di normale buon senso, accolta molto positivamente dal relatore Astorre, che ringrazio. Mi riferisco all'obbligo per tutti gli scuolabus di dotarsi di cinture di sicurezza per gli studenti entro la fine di quest'anno; agli incentivi per il conseguimento della patente per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e merci; alla destinazione delle risorse per l'assunzione di nuovo personale qualificato presso le motorizzazioni civili, per sopperire alla carenza di organico ormai decennale. Mi riferisco - e ringrazio particolarmente la collega, senatrice Saponara, per la proposta che io da montanaro vivo e sento particolarmente - all'ordine del giorno che prevede l'estensione della misura Resto al Sud, oltre che alle isole minori, lagunari e ai Comuni insulari, anche ai Comuni montani: una sorta di "Resto in montagna" per prevenire la desertificazione. Questo non è poca cosa, almeno negli intenti. Mi riferisco al reperimento delle risorse per l'avvio dei lavori sulle funivie di Savona, che il collega Ripamonti perora da diverso tempo, e allo sblocco del progetto della tangenziale di Demonte e allo stanziamento di risorse destinate alla realizzazione della variante tra Pieve di Teco e Ormea e alla messa in sicurezza della strada statale 28. Sono tutte proposte di buon senso che arrivano dal territorio e che ci fa piacere siano state accolte in Commissione. Questi ordini del giorno arricchiscono il provvedimento e stimolano molti altri interventi a favore dei cittadini; mi congratulo, quindi, con il Governo per averli presi in considerazione e ringrazio tutti i colleghi che in Commissione li hanno sostenuti, benché il tempo sia stato veramente molto limitato. Ora attendiamo fiduciosi che questi ordini del giorno si trasformino in atti concreti da parte del Governo, cui seguiranno ovviamente ulteriori proposte della Lega. al testo del decreto-legge in esame, tutti i provvedimenti sono ovviamente perfettibili. In tema di monopattini elettrici esprimiamo rammarico per quella che, a nostro giudizio, è un'occasione mancata. Nonostante alcune novità positive introdotte in Commissione alla Camera, grazie al contributo della Lega, come ad esempio il divieto di transito e sosta sui marciapiedi per questi monopattini, nonché la riduzione da 25 a 20 chilometri orari della velocità, la previsione di confisca in caso di modifiche che ne aumentino le prestazioni, purtroppo molti altri nodi sul fronte della sicurezza stradale sono ancora aperti, soprattutto con riferimento alla obbligatorietà del casco e alla questione delle targhe e delle assicurazioni. Grazie alla Lega siamo entrati nel merito di alcune scelte sui monopattini e sulle auto elettriche, di alcune problematiche della motorizzazione, degli estremi disagi che ci sono in questo Paese. Avremmo sperato che il Governo osasse di più con questo decreto-legge. Rimaniamo tuttavia fiduciosi che si possa in futuro fare meglio e rimarremo sempre proattivi su questi temi. Abbiamo comunque avuto successo sui temi del lavoro portuale, delle infrastrutture, della vocazione marittima del nostro Paese. Abbiamo reperito fondi e investimenti e siamo riusciti anche a semplificare opere pubbliche, come la diga di Genova, a rivedere questioni che erano ferme, come la autostrada A22 e le opere olimpiche, che finalmente saranno avviate. In merito alla A22, già citata ieri dal presidente Coltorti, ribadisco l'importanza dell'opera come prolungamento naturale della bretella Sassuolo-Campogalliano; quest'opera è il vero banco di prova per quella buona politica in cui tutti gli imprenditori e gli operatori, non sono del comparto ceramico, ma anche di quello biomedicale, del turismo, del tessile, della meccanica, dell'agricoltura, credono ancora. È evidente che è stato fatto un grande lavoro di collaborazione tra tutte le componenti della maggioranza di questo Governo, almeno in Commissione, nel poco tempo a disposizione; ma è altrettanto evidente che non possiamo più far attendere queste opere di primaria e strategica importanza, cui speriamo si aggiungono a breve molte altre. Mi permetto di sottolineare l'egregio lavoro svolto in brevissimo tempo dai componenti dell'8a Commissione, dal presidente Coltorti e dal relatore senatore Astorre, che ringrazio.

hanno avuto l'onore di dare un contributo e di migliorare questo decreto-legge, visto che a noi non è stato concesso. Purtroppo i tempi lunghi dei lavori alla Camera hanno contratto i nostri tempi e questa volta ne abbiamo sofferto noi, che siamo i senatori della Repubblica. A questo oggi si aggiunge anche la questione di fiducia posta dal Governo. Governo. Credo che, anche ascoltando tutti gli interventi dei nostri colleghi, possiamo dire che il tema più largamente condiviso è proprio è proprio quello dell'insofferenza dei Gruppi rispetto a queste dinamiche. *(Applausi)*. Per questo vorrei scuotere il Governo, affinché ci renda più partecipi nella gestione e nelle dinamiche dei provvedimenti.

prevedevano solo ed esclusivamente un rafforzamento della sicurezza nella circolazione stradale, introducendo il cosiddetto codice rosa. Tuttavia, durante i lavori alla Camera, ci sono state numerose modifiche. Principalmente, voglio ricordare la modifica apportata all'articolo 1 del codice della strada, dove viene inserita per la prima volta la parola ambiente, che credo sia espressione cosa molto *in auge* in questi giorni.

Sembra una cosa da niente, ma non lo è, se pensiamo che la tutela e l'attenzione all'ambiente, oggi più che mai, devono avere una corsia preferenziale da percorrere. Come legislatori, noi abbiamo l'obbligo morale di perseguire questo fine e di raggiungere gli obiettivi che il Paese, l'Europa e il mondo intero si sono dati. È per questo che, come MoVimento 5 Stelle, possiamo riconoscere l'avvio di un percorso che ormai stiamo tracciando e che, colleghi, stiamo tracciando insieme. Di questo non possiamo che essere felici e registrare la differenza nel modo in cui ci guardate. Non ci guardate più con quell'ambiguità

una priorità importante, che è proprio quella dell'ambiente che è nel nostro simbolo. C'è dell'altro in questo decreto. In particolare, vi è un tratto davvero innovativo per il nostro Paese, che ci avvicinerà, in termini di sensibilità ambientale e faunistica, ad altri Paesi decisamente più avanzati di noi in questo ambito. Sto parlando dell'obbligo di prevedere, durante la fase di progettazione di nuove opere stradali, autostradali e ferroviarie, infrastrutture complementari chiamate corridoi verdi; delle infrastrutture che saranno utili a consentire il passaggio in sicurezza della fauna selvatica. Mi auguro che, quanto prima, questa visione possa essere ulteriormente ampliata e possa permettere di prevedere la realizzazione di veri e propri ecodotti anche sulle infrastrutture già esistenti. Non è possibile, infatti, che oggi, nel 2021, siamo costretti ancora a leggere notizie che riportano le morti di animali selvatici come cervi o addirittura orsi, quindi specie protette, perché non riusciamo ad arginare la loro introduzione sulle carreggiate delle nostre infrastrutture stradali e autostradali. È un fenomeno lontano anni luce da quello che l'Unione europea si è prefissato come obiettivo strategico, ovvero quello di dimezzare il numero dei feriti gravi entro il 2030 e di azzerarlo entro

Sembra strano ed illogico, ma oggi parliamo ancora di questo. Registriamo, però, un passo avanti anche se, come MoVimento 5 Stelle, vogliamo puntare a molto di più. Così come risulta incredibile ancora oggi che i piani economico-finanziari delle concessioni autostradali siano oggetto di ulteriori proroghe. Signori del Governo, dobbiamo dircelo chiaramente. Dobbiamo essere chiari con i nostri elettori, dobbiamo essere chiari con i cittadini e dobbiamo essere chiari anche con noi stessi: ci sono concessioni che non sono in ritardo di mesi, ma di anni. La rimodulazione dei piani di gestione permetterebbe di applicare quel nuovo sistema

Io vorrei dire basta a queste proroghe e andiamo avanti con l'applicazione delle norme, che esistono e ridanno un senso e un equilibro ai rapporti tra Stato e privato, a favore dello Stato e del cittadino naturalmente. Poi c'è la questione della *Newco* interamente controllata dal MEF, soggetta a controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Si prevede che ad essa vengano trasferite tutte le funzioni che ad oggi sono attribuite ad ANAS, con l'esclusivo riguardo delle autostrade statali a pedaggio. Io ritengo che questa è un'ottima soluzione; una soluzione che va nella giusta direzione, ovvero quella del ritorno delle concessioni nelle mani dello Stato. parere, se questa soluzione fosse stata attuata prima, allora ci saremmo evitati di leggere nel decreto delle soluzioni ambigue come quella trovata per la A22 (la

dovremmo acquisire un parere del Governo relativamente ad eventuali profili di incompatibilità di questa norma con quella europea in materia, perché ricordiamo che è notizia di pochi mesi fa di una lettera pervenuta all'Italia da parte della Commissione europea in cui c'era la comunicazione della messa in mora dell'Italia al fine di garantire la corretta attuazione delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione. Secondo il diritto dell'Unione europea, infatti, la proroga di una concessione equivale a una nuova concessione e può essere aggiudicata solo mediante una procedura di gara. Sarebbe paradossale ricevere da Bruxelles un deferimento alla Corte di giustizia europea, uno scenario che questo Governo, come qualunque altro Governo, dovrebbe evitare. Tornando al codice della strada,

di tentativi di convergenze con gli altri gruppi politici non si siano persi nel nulla. Fortunatamente, non è stato questo il caso, come non è stato il caso di mandare in fumo investimenti di un intero settore, cioè quello della micromobilità elettrica comunemente definita nell'ambito dei monopattini. Colleghi, quante volte vi abbiamo sentito fare battute, rilasciare interviste attraverso le quali si tentava di demonizzare questi innovativi strumenti? Molti l'hanno definita una stretta sul settore, quella che è contenuta in questo decreto, invece dobbiamo essere nuovamente onesti, ma dobbiamo esserlo tutti e dire che al contrario si tratta di una stretta necessaria che salva l'esistenza e la circolazione dei mezzi di micromobilità nelle nostre città. Si è evitato di lasciare tanti cittadini senza una parte fondamentale della mobilità urbana e ricordiamo apertamente che la vera stretta sarebbe stata quella di imporre l'obbligo del casco a tutti, quando invece è stato imposto solo ai minori ed in virtù della loro sicurezza personale; imporre l'obbligo dell'assicurazione e della targa o addirittura il divieto di circolazione di questi mezzi nelle ore serali ai minorenni. Su questo e sulla delicata questione per noi fondamentale delle concessioni autostradali, non ci fermeremo e continueremo a lavorare e se necessario anche a dare battaglia. Resta il fatto che in questo provvedimento mettiamo al loro posto tanti tasselli, tutti importantissimi ed è questa la politica che gli italiani oggi ci chiedono in questo frangente. Dichiaro pertanto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

voglio partire da un punto molto semplice, che non interessa forse nessuno, quindi potete continuare a parlare, cioè che avevo dato la fiducia a questo Governo a suo tempo. la fiducia di una sola persona, di un solo parlamentare, quando il Governo ha circa il 90 per cento del sostegno parlamentare, è del tutto irrilevante e allora non parlo in termini politici di sostegno al Governo, ma in termini giuridici. Ho sentito quasi tutti i miei colleghi che sono intervenuti lamentare il fatto che il Governo ci ha lasciato meno di quarantotto ore di tempo per esaminare un provvedimento *omnibus* a senso unico alternato, come si dovrebbe dire, che svuota il Parlamento e ci si lamenta nei confronti del Governo. Si chiede al Governo di rispettare il Parlamento.

Tendete le mani, ma non per soccorrere qualcuno dal mare, voi tendete le mani perché il Governo ci lasci qualcosa. Questa è la verità, perché voi non avete il coraggio e la dignità di pretendere il rispetto del Governo. In questo provvedimento - l'avete detto tutti - non sappiamo cosa ci sia esattamente. Abbiamo letto i titoli e vi sono stati annunciati. La verità è che qui dentro c'è lo scardinamento del diritto del lavoratore, c'è lo scardinamento delle relazioni sindacali. Anche se qualcheduno alza la voce e critica, non ha poi il coraggio di essere coerente e conseguente.

Questo è un provvedimento illegittimo che svuota il Parlamento, in quanto è un decreto *omnibus* (il Presidente della Repubblica l'ha detto più volte). secondo luogo, è viziato, perché alla base dell'articolo 7 c'è un atto segreto: è inammissibile e inaccettabile, in democrazia, che si converta in legge un provvedimento sulla base di un atto segreto.

strumenti e uomini, però in questo caso no: passano soltanto i capitali, gli *asset* e i bulloni, ma gli uomini e i contratti; i lavoratori sono lasciati soli e nudi davanti all'imprenditore padrone,

n. 121, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: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 votazione nominale con appello. Ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti (che si sono già costituiti prima ancora di partire). Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della giustizia.

*(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, il decreto-legge in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi ha previsto già nel 2019, nell'ambito del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, uno stanziamento di 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sostenere la rigenerazione della olivicoltura, che in Puglia è stata - come sappiamo - infetta da xylella fastidiosa. In attuazione di questo disposto, il decreto del Ministro delle politiche agricole del 6 marzo 20, di concerto con il Ministro del Sud e della coesione e con il Mise, ha previsto la ripartizione dei 300 milioni di euro complessivi ed istituito, per garantire piena attuazione del piano straordinario, un comitato di sorveglianza, prevedendo le sue riunioni con cadenza almeno semestrale. Diverse disposizioni del citato decreto ministeriale stabiliscono le funzioni cui è chiamato il comitato di sorveglianza. Tra le numerose, mi piace richiamare richiamare la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per gli importanti interventi, quali, innanzitutto, la rimozione delle piante disseccate e infette a causa della xylella o il reimpianto degli ulivi, sempre nelle zone infette, o ancora la riconversione verso altre culture. Con un comunicato del 30 aprile 2020 il Ministero ha annunciato l'insediamento del comitato di sorveglianza. Ora, a distanza di un anno e mezzo, molti attribuiscono alla mancata convocazione dello stesso comitato la responsabilità di aver congelato lo stanziamento delle risorse per i numerosi progetti già predisposti. Trovo ultroneo ribadire che, per la completa attuazione di quel piano straordinario, è per noi elemento dirimente l'effettivo impiego delle risorse stanziate. Anzi, bisognerebbe aggiungerne delle altre. Io intendo chiedere al signor Ministro quali iniziative intenda assumere per assicurare la effettiva erogazione delle risorse e se il Ministero abbia fatto tutto quello che era nelle sue possibilità, giacché, anche nelle audizioni fatte in Regione nelle ultime settimane, è stato affermato che è colpa del Dicastero non aver osservato i tempi e gli adempimenti. PRESIDENTE. Il Ministro

già con decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, è stato approvato il piano di riparto dei 300 milioni di euro per la rigenerazione olivicola della Puglia sono stati istituiti un tavolo di coordinamento emergenza xylella, con il compito di valutare l'attuazione dell'intero piano e decidere l'allocazione delle risorse tra le diverse misure, e un comitato di sorveglianza, istituito con decreto ministeriale nell' aprile 2020, con il compito di esaminare i singoli provvedimenti attuativi. Occorre rilevare che, a differenza del tavolo di coordinamento, il comitato di sorveglianza si è riunito il 30 aprile 2020, il 22 maggio 2020, il 18 febbraio 2021 ed è stato consultato anche in data 19 giugno 2020. Il piano di riparto ha previsto diverse allocazioni. Tre sono le misure principali, poi vi è una serie di misure più piccole, da pochi milioni di euro. La misura principale è il sostegno reddito, 120 milioni di euro che sono stati interamente ripeto, interamente - erogati dal Ministero alla Regione Puglia. Quanto allo stato di attuazione, però, non disponiamo di informazioni rispetto alle risorse effettivamente trasferite alle imprese danneggiate. Per quanto riguarda la misura che prevede il reimpianto di ulivi in zona infetta, vi è un intervento fondamentale da 40 milioni di euro. Per questa misura, sappiamo che - come comunicatoci il 25 ottobre 2021 dalla Regione Puglia - sono state presentate complessivamente 8.133 domande; richieste di espianto di 3,8 milioni di alberi su 31.900 ettari, con un fabbisogno complessivo di circa 222 milioni, ma non abbiamo maggiore contezza rispetto alle motivazioni delle richieste delle singole aziende. La terza misura di rilievo è quella da 25 milioni di euro per la riconversione verso altre colture. La lista delle specie resistenti a xylella è stata da poco approvata dal Comitato fitosanitario nazionale e il relativo provvedimento è in fase di adozione rispetto alle risultanze del Comitato stesso. Ciò premesso, abbiamo convocato

questo, ci sono 100 milioni nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nella procedura di meccanizzazione destinata al tema dell'olio d'oliva, e quindi a supporto dei territori che lo producono, e ieri è stato dato dalla Conferenza Stato-Regioni il concerto sul decreto da 30 milioni che riguarda sempre

è su due fronti: quello di essere severo nell'attuazione delle procedure, perché il territorio è mortificato e devastato da questo patogeno e abbiamo la necessità di riconvertire, di ricominciare; le iniziative appena citate del Governo, attraverso le quali rifinanziare con nuove risorse ulteriori progetti. Parliamo di un fenomeno enorme, e lo ha detto bene lei: a fronte di 20 milioni di euro disponibili, con 8.281 domande di reimpianto la richiesta supera i 220 milioni. Abbiamo necessità di dare risposta agli agricoltori, ai proprietari dei nostri oliveti pugliesi, perché non possiamo tradirli doppiamente

*(L-SP-PSd'Az)*. Signor Ministro, ancora una volta siamo in quest'Aula a chiedere l'attenzione sua e del Governo a difesa della dieta mediterranea e, su tutto, per combattere la ormai troppo invasiva comunicazione per cui la carne sintetica sarebbe migliore di quella proveniente dalla nostra zootecnia nazionale. Sono ormai due anni che EAT-Lancet Commission ha pubblicato un *report* nel quale viene delineata una strategia per un'alimentazione universale, andando nei fatti a omologare le scelte dei consumatori. Tali posizioni integraliste stanno influenzando anche gli orientamenti della Commissione europea sulla transizione ecologica, la quale pare stia finanziando, con i soldi della ripresa economica post-Covid, la ricerca sui cibi sintetici. Non vogliamo essere complottisti, ma molti organi di informazione riportano di oltre due milioni di euro concessi a multinazionali olandesi sostenute da fondi in cui hanno investito anche attori, magnati dell'informatica, dei *social* e dello sport. ormai in atto un'evidente strategia per screditare il *made in Italy* a favore di modelli alimentari assolutamente lontani dalla nostra cultura, dalla tradizione, dalla stagionalità che sono basati sulla promozione di cibi ultraprocessati e sintetici che vengono promossi senza aver verificato le conseguenze. E questo è gravissimo. Occorre pretendere dai regolatori europei e da quelli nazionali la massima rigidità nel valutare gli effetti di questi prodotti sintetici anche a lungo termine sulla salute e sulla dieta dei nostri consumatori. Queste posizioni indeboliscono poi le filiere e la competitività delle filiere agroalimentari italiane, già duramente provate dall'emergenza sanitaria, con lo *stop* alla ristorazione e il calo delle vendite e dei prezzi, a cominciare dal settore zootecnico, che conta - lei lo sa - 115.000 aziende attive nel nostro Paese, 250.000 occupati e un patrimonio di 17 miliardi di euro (80 miliardi si valuta il giro d'affari al consumo). Ad avvantaggiarsene sono le multinazionali del cibo, che stanno investendo in tecnologie innovative per produrre carni sintetiche. Il tentativo è insinuare nell'opinione pubblica che la carne rossa danneggi la salute dei consumatori, che gli animali negli allevamenti siano maltrattati e che la zootecnia produca spreco di acqua e generi un'elevata emissione di anidride carbonica. Questa non è la visione reale. In Italia gli allevamenti hanno adottato tecniche di produzione a basso impatto ambientale, con un'attenzione particolare al benessere animale. Noi le vogliamo chiedere, signor Ministro, che cosa intende fare, in questo momento di grave difficoltà, per rendere competitiva la zootecnia, anche attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, soprattutto perché la transizione ecologica deve diventare un motivo non per favorire carne sintetica, il pesce sintetico o qualsiasi altra roba sintetica, ma per investire in politiche attive mirate alla crescita sostenibile delle filiere agroalimentari italiane, a difesa della salute e della libertà di scelta dei consumatori. *(Applausi)*.

ho ripensato al film «Matrix» - penso che tutti voi lo ve lo ricordiate bene - quando il gruppo di Morpheus si accorge che la realtà in cui viviamo è virtuale e si cala nel mondo reale, dove gli uomini sono delle batterie attaccate con un cavo. Per sopravvivere in quel mondo devono mangiare una pappa piena di proteine, vitamine, eccetera; un nutriente senza gusto, prodotto in modo sintetico. Se c'è qualcuno che pensa che quello sia il modello di riferimento a cui dobbiamo portare il mondo intero, con sistemi alimentari prodotti in laboratorio e nelle fabbriche,

non deve essere confusa con la strategia *one diet*, perché non esiste una dieta unica che vada bene per ciascun essere umano. E non esiste un cibo buono che fa bene e un cibo insano che fa male. Esistono diete equilibrate. Gli eccessi fanno male, ma il consumo equilibrato di proteine animali, di proteine vegetali e di tutti i tipi di nutrienti è l'unico modo che abbiamo per fare una vita sana, magari accompagnata da un po' di attività sportiva. è chiaro che il settore della zootecnia, oltre a questi attacchi, presenta anche delle criticità legate alla revisione della nuova PAC; sappiamo benissimo che i percorsi di convergenza interna porteranno a una riduzione degli interventi a favore della zootecnia. È proprio per questo che stiamo costruendo, nella nuova PAC e nel Piano strategico nazionale,

di far vedere quanto di buono quella filiera ha fatto, affidando all'organismo di certificazione la verifica del rispetto dell'impegno di pascolamento. Ma non c'è soltanto questo. Nella legge di bilancio abbiamo riproposto la norma sulla compensazione IVA, che vale 74,5 miliardi nel settore della zootecnia. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza cerchiamo di accompagnare la resistenza di reddito della zootecnia attraverso misure complementari, come il passaggio al biogas e al biometano, che è molto importante per il settore zootecnico, o come la misura agrisolare, che consentirà un'indipendenza energetica a quelle aziende. Quindi, ci sono risorse sia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che nella legge di bilancio, ma soprattutto il Governo, il Parlamento

Signor Presidente, ringrazio il ministro Patuanelli. Noi della Lega siamo convinti che lei stia facendo tutto il possibile per la difesa del *made in Italy* e soprattutto della dieta mediterranea

perché è notizia di circa due mesi fa che l'Unione europea ha approvato la farina di larve e, quindi, gli insetti come cibo. Assolutamente non vogliamo che ciò vada in porto. Sappiamo che la dieta mediterranea è famosa in tutto il mondo; è patrimonio immateriale dell'umanità e la controprova ne è il fatto che l'Italia è sicuramente in Europa il Paese più longevo. Se viviamo più degli altri, significa che mangiamo bene. Oggi è una giornata sicuramente suggestiva: il 4 novembre

Le nostre stalle stanno soffrendo; il prezzo del latte è sicuramente un punto su cui dobbiamo porre più attenzione e poi ricordiamoci tutti la questione delle quote latte. In questo momento le stalle stanno chiudendo.

Signor Presidente, onorevole Ministro, il prezzo delle materie prime è salito nella maggior parte dei settori industriali per ragioni logistiche e speculative. Ciò è dimostrato dal prezzo della macro categoria delle terre rare. Di preciso, il valore del rodio è aumentato del 447 per cento e ciò ha creato un fenomeno che gli economisti inglesi hanno soprannominato *everything* *bubble*. Premesso che l'incremento del prezzo è accompagnato dalla mancata disponibilità sul mercato, causata dalla simultanea ripartenza produttiva di tutto il mondo dopo l'interruzione che c'è stata con l'emergenza Covid; premesso che l'economia italiana dipende in gran parte dall'importazione di materie per sostenere le proprie aziende, come è stato dimostrato dall'Istat nel documento Ecomondo 2020, in cui si stima che la somma del valore complessivo delle importazioni di materie prime si aggira intorno ai 18,6 miliardi di euro; considerato che l'indisponibilità di *slot* all'interno dei *container* marittimi, accompagnata da un aumento dei prezzi del trasporto, ha causato ingenti danni all'impresa italiana, con la conseguenza che molte commesse sono state attivate con contratti che hanno previsto delle penali per mancata consegna e che da alcune settimane si susseguono conseguentemente segnalazioni di carenze di materie prime da tante categorie di industria, artigianato e produzione; considerato che è fondamentale garantire che le filiere di molti settori non vengano interrotte per la carenza di componentistiche che potrebbero comportare la sosta di importanti aziende nel settore della meccanica e dell'edilizia; considerato che una situazione di questo tipo può determinare conseguenze negative per il PIL e, quindi, per i posti di lavoro e considerando anche che si può sospettare che, proprio per i motivi succitati, i mercati delle materie prime possono essere oggetto di azioni speculative, pensiamo che il problema logistico marittimo abbia sicuramente influenzato i prezzi delle materie prime provenienti dall'Oriente, dall'Africa del Nord, dagli Stati Uniti, dal Nord e dal Sud dell'America e, quindi, pensiamo che per aiutare le imprese italiane sia importante rafforzare gli scambi con i *partner* europei. Per questo motivo chiediamo al Ministro, che è sicuramente a conoscenza di queste situazioni, che

Signor Presidente, onorevoli senatori, nel corso degli ultimi mesi è emersa una grande preoccupazione per l'aumento globale dei prezzi delle materie prime, per le imprese e per le famiglie. Le cause che caratterizzano questo fenomeno sono diverse, a seconda della tipologia di bene e di settore: si va infatti da tematiche geopolitiche a fenomeni meramente speculativi, con un dato ormai caratterizzante, che è rappresentato da un rapporto tra domanda e offerta che ha spinto i prezzi al rialzo. Si tratta in parte di fenomeni contingenti, motivati da picchi di domanda o da transitorie carenze di specifiche materie prime, ma il rischio di essere solo all'inizio di una fase di generale rincaro dei prezzi non è certo trascurabile. Di fronte a queste evidenze, occorre interrogarsi in primo luogo sugli strumenti a disposizioni per contrastare il fenomeno. In determinati casi, come nel settore dell'energia, si è intervenuti con specifiche disposizioni a livello nazionale: faccio riferimento al decreto-legge n. 130 del 2021, con il quale sono state adottate misure specifiche di contenimento dei prezzi nel settore energetico e del gas naturale. Si tratta tuttavia di interventi contingenti, a cui si devono affiancare misure più strutturali di lungo periodo, a carattere necessariamente strutturale, come anche di recente ribadito dal presidente del Consiglio, Draghi, con la necessità di una strategia a livello europeo che punti all'autonomia strategica dell'Unione su su diversi temi, a partire dell'energia: di questo si è parlato recentemente nei *summit* che si sono tenuti a Roma. In altri settori, come quello dell'acciaio, uno dei nodi principali è costituito dal sistema di quote e dazi previsto dalla Commissione europea, variabile a seconda dei Paesi di importazione, inizialmente introdotti per tutelare gli interessi delle aziende europee, ma che allo stato rischiano di produrre un effetto dirompente, a cui occorrerà far fronte a livello di Unione europea, mediante un rapido ripensamento degli attuali limiti. probabilmente si potrà parlare, anche alla luce delle recenti dichiarazioni venute dalla controparte statunitense. Per altre materie prime il discorso è ancora più complesso: si pensi al rame, la cui domanda ha subito un'impennata, visti i settori ove il suo impiego è cruciale. Vi sono poi casi in cui l'aumento dei prezzi è almeno parzialmente l'effetto di politiche di incentivazione nazionale, come - ad esempio - nel settore dell'edilizia, dove i *bonus* hanno determinato quello che può essere definito un vero e proprio effetto *doping*, che, sommato alla carenza a livello globale di determinate materie prime, ha determinato oggettive criticità. In questo contesto, la rimodulazione del sistema incentivante e la ridefinizione di un adeguato sistema di prezziari sono interventi che, a livello governativo, appaiono necessari, ma che possono solo in parte arginare il fenomeno, che in questo caso assume comunque un carattere per lo più contingente. *(Richiami del Presidente).* Nota a tutti è poi la carenza di offerta dei semiconduttori, che non ha determinato solo un innalzamento dei prezzi, ma anche una vera e propria criticità a livello mondiale, che ha rallentato o bloccato intere filiere produttive. A livello europeo l'attenzione al tema dell'aumento dei prezzi è comunque altissima. Il Piano di azione sulle materie prime critiche è stato progressivamente ampliato e nella sua ultima versione, risalente però a settembre 2020, è stata aggiornata la lista di materie prime critiche ed è stato formulato un rapporto prospettico. si sviluppa su diverse linee di azione e mira: a sviluppare catene del valore resilienti per gli ecosistemi industriali dell'Unione europea; a ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche primarie mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione; rafforzare l'approvvigionamento interno di materie prime dell'Unione europea; a diversificare l'approvvigionamento dai Paesi terzi e rimuovere le distorsioni del commercio internazionale. Sono tutte materie che - lo ricordo

A tal fine, oltre all'utilizzo degli strumenti a disposizione dei Governi nazionali, è necessario promuovere un quadro europeo di interventi unitario, finalizzato a iniziative e soluzioni armonizzate, per garantire l'approvvigionamento di materie prime, materiali e prodotti di base e sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese.

il Gruppo Fratelli d'Italia è molto preoccupato per gli sviluppi che sono seguiti alla grave crisi dell'Alitalia. Nel corso degli anni la Compagnia ha rappresentato un biglietto da visita del nostro Paese per il settore dei trasporti e per tutte le nostre eccellenze. Una compagnia aerea nazionale importante è fondamentale per i grandi Paesi come il nostro, in particolare quando si è una Nazione che vede nel turismo una delle sue risorse principali e quella con

nel corso degli anni Alitalia ha assorbito molto denaro, in parte denaro pubblico, in parte denaro privato,

Per anni si era detto che i dipendenti di Alitalia guadagnavano più dei loro colleghi stranieri, anche se spesso non era vero, ma adesso è diventato vero il contrario, nel senso che guadagnano di meno e hanno condizioni lavorative più difficili. e il protrarsi della crisi più volte Fratelli d'Italia ha presentato delle proposte. Nel giugno scorso abbiamo presentato delle proposte concrete una mozione che si preoccupava dei vari settori in cui era possibile intervenire. Noi oggi le chiediamo, signor Ministro, quali sono le

quali sono le prospettive del trasporto. Abbiamo chiesto, e tuttora auspichiamo, un coordinamento tra le modalità aerea, ferroviaria, portuale e viaria. È necessario compiere un grande lavoro in questo senso, grande lavoro in questo senso, facendo in modo che delle aziende nascano, si sviluppino o abbiano l'assetto adatto ad affrontare le emergenze di questi anni in tutto il settore di supporto, con l'indotto che può essere quello di una grande compagnia aerea.

come Ministro dello sviluppo economico anche se, come sapete, ITA è una compagnia aerea posseduta al 100 cento dal MEF e, quindi, il piano industriale fa riferimento a quel Ministero.

sempre consentite in termini di discontinuità aziendale. La parola chiave, in tutto questo processo molto complicato che prevede - appunto - il rispetto sia della normativa europea sia delle normative nazionali per quanto riguarda le procedure di cui alle leggi Prodi e Marzano, deve rispondere a tale criterio. È questo il motivo per cui l'azionista è il MEF e gli organi si stanno muovendo con una discontinuità che è andata anche a incidere sul contratto di lavoro che è stato adottato e che risponde esattamente a una delle prescrizioni fatte dalla Commissione europea. Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, il Governo si è mosso subito assicurando un sistema di ammortizzatori sociali che dovrebbe accompagnare il piano di sviluppo aziendale, piano di sviluppo aziendale, che parte in condizioni oggettivamente di perimetro limitato, ma che dovrebbe assorbire - ovviamente se il mercato ci assisterà - migliaia di lavoratori già a partire dall'anno prossimo, fino ad arrivare possibilmente nell'orizzonte pluriennale per quanto riguarda l'*handling* e la manutenzione, in questo caso si va verso gare a cui sicuramente l'auspicio è che ITA, in concorrenza e in cooperazione con investitori privati,

vedere un sistema integrato tra il viaggio aereo e le ferrovie. È, quindi, questo un obiettivo di sistema che assolutamente vogliamo perseguire. È altrettanto evidente che il successo dell'operazione di ITA di ITA deve darci forza e capacità negoziale, perché nel futuro mercato del settore aereo anche l'interlocuzione con altri vettori, in vista di alleanze strategiche, richiede di andare al tavolo a testa alta e con i conti in regola.

anche a tutta la struttura aeroportuale del nostro Paese non può che trovarci d'accordo. Certo, per ora vediamo anche grandi criticità,

È importante non soltanto per i dipendenti di Alitalia, non soltanto per l'indotto, che pure ha la sua grande rilevanza, ma anche per tutto il Paese avere una compagnia che abbia il suo peso, che eviti alla maggior parte dei viaggiatori di fare

Paesi dove comunque devono transitare. È importante che il Governo e l'Italia nel suo insieme facciano pesare anche in sede internazionale l'importanza che ha per noi avere una compagnia, un trasporto aereo che sia attraente per gli investimenti, per il turismo e che naturalmente serva adeguatamente anche all'interno dell'Italia. Su questo noi saremo sempre pienamente collaborativi e speriamo che il Governo faccia valere tutto il peso del nostro Paese in questo senso.

Signor Presidente, Ministro, un terremoto ha di recente sconvolto il mondo dorato delle ditte che forniscono a detenuti e internati il vitto e il sopravvitto. Vitto è il cibo necessario al confezionamento dei tre pasti giornalieri assicurati dall'amministrazione attingendo alla diaria *pro capite* di ciascun ristretto; extravitto o sopravvitto sono i generi alimentari e di conforto che invece si acquistano a piacere, ma con denaro proprio. Ai primi di settembre la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con le delibere nn. 101, 102, 103 e 104 del 2021, ha negato il visto e la registrazione dei decreti di approvazione di altrettanti contratti predisposti dal DAP tramite il provveditorato regionale di Lazio, Abruzzo e Molise, contratti di fornitura del vitto per il triennio 2021-2023 negli istituti di Rebibbia per quasi 4,5 milioni di euro, di Civitavecchia e Viterbo per 2,2 milioni, di Abruzzo e Molise per 2,5 milioni, di Frosinone, Cassino e Latina per 1,7 milioni. Benché nel 2020 la base d'asta sia stata aumentata da 3,90 a 5,70 euro giornalieri e la media nazionale si aggiri sui 3,92 euro, le offerte delle tre imprese che si erano aggiudicate i quattro contratti, poi annullati in autotutela, riferite in base alla *lex specialis* di gara solo al servizio principale e obbligatorio di vitto, prevedevano ribassi vicini o addirittura superiori al 60 cento: 2,39 euro giornalieri *pro capite* la ditta Domenico Ventura srl e addirittura 2,25 euro la ditta Ragionier Pietro Guarnieri-figli srl, mentre la Sirio srl ha proposto 3 euro. Di qui - osserva la Corte - l'apparente insostenibilità economica del servizio di vitto, ove svincolato dai ricavi del sopravvitto, e l'evidente detrimento del principio di qualità delle prestazioni. Anzi, con il presidente Antonio Mezzera, il collegio di controllo preventivo non solo ha segnalato l'anomalia dello straordinario ribasso con cui vengono affidati tali contratti di fornitura di vitto giornaliero completo, circostanza difficilmente compatibile con una dignitosa alimentazione della popolazione carceraria, ma ha stigmatizzato che per un appalto e una concessione di servizi sia bandita un'unica procedura invece di due. La pronuncia del Consiglio di Stato lo scorso agosto e poi quelle della Corte dei conti di fatto confermano le denunce raccolte, ad esempio, dal Garante dei detenuti di Roma, Gabriella Stramaccioni, circa l'insufficienza del vitto e i costi esorbitanti del sopravvitto a Rebibbia e ha sollecitato la stampa più attenta a puntare i riflettori su questa prassi francamente scandalosa. Poiché non è accettabile sul piano etico e non è consentito lucrare sulla pelle dei detenuti, si chiede al Ministro interrogato di quali informazioni sia in possesso al riguardo e quali iniziative intenda assumere per garantire ai detenuti negli istituti di pena i basilari principi umanitari desumibili degli articoli 27 e 32 della Costituzione,

Presidente, il problema che è posto alla nostra attenzione è quello del vitto e del sopravvitto nelle carceri. Distinguerei due profili dell'interrogazione che è stata presentata, peraltro connessi fra di loro: uno è quello giuridico, messo in rilievo dalle pronunce della Corte dei conti e del Consiglio di Stato nei bandi di gara, in particolare per quanto riguarda il provveditorato del Lazio e Regioni limitrofe, e l'altro, che è accennato nel finale, è relativo relativo alla scarsa qualità del cibo denunciato da alcuni organi di stampa e che va a detrimento, evidentemente, della dignità dei detenuti. Sul primo profilo, i problemi giuridici legati ai bandi e alle gare del vitto e del sopravvitto sono all'attenzione dell'amministrazione penitenziaria da tempo, in particolare da quando, nel 2017, sono entrati in vigore dei principi dell'Unione europea che superano le procedure negoziate fra l'amministrazione e le parti a favore di un'apertura al mercato comune. Ci sono state gare bandite nel 2017 e annullate dal Consiglio di Stato per una base d'asta ritenuta troppo bassa, poi l'amministrazione ha dato indicazioni diverse e sono state rifatte delle gare nel giugno 2020, anche se poi nuovamente annullate. Insomma, il tema della corretta erogazione del vitto e del sopravvitto è all'attenzione dell'amministrazione penitenziaria, soprattutto a seguito delle pronunce del Consiglio di Stato del 2021 e della Corte dei conti,

in una delle pronunce da lei citate, la mancata separazione espone al rischio di «improprie compensazioni, da parte delle imprese, tra i minori costi del vitto (praticati per ottenere l'affidamento del servizio) e i maggior introiti ricavabili dal sopravvitto a discapito della qualità dei servizi alimentari primari offerti ai detenuti». Dunque, questo è un punto cruciale: bisogna operare una doverosa separazione dei servizi e delle procedure. Il bando del Lazio, che è stato rifatto, ha mantenuto una base d'asta superiore. C'è tanto lavoro da fare. Vedo che il tempo a disposizione sta già per scadere. Segnalo soltanto che, da un lato, la competenza per i bandi del vitto e sopravvitto è dei provveditorati e non dell'amministrazione centrale; la qualità, il controllo del sopravvitto è affidato ai regolamenti interni di ciascun istituto penitenziario. il 13 settembre ho convocato una commissione per l'innovazione del sistema penitenziario che, proprio su questo punto, è subito intervenuta dando tre indicazioni. La prima è che sempre nella predisposizione, le procedure di aggiudicazione del vitto e sopravvitto debbono essere distinte: contratto d'appalto del servizio del vitto e contratto di concessione per il sopravvitto. è che devono essere escluse le rimodulazioni del minimo al ribasso; la terza è che occorre, nella costruzione della qualità dei prodotti offerti, un parere obbligatorio e vincolante da parte di un tecnologo alimentare per le caratteristiche nutritive e qualitative di ogni prodotto previsto nel capitolato contenuto in un decreto ministeriale.

per la puntualità con cui ha ricostruito la fornitura di vitto ed extra vitto nei penitenziari italiani, in particolare dando risalto alla svolta del 2017, alla quale - possiamo dircelo - l'associazione degli appaltatori dei contratti in questione non si è ancora assuefatta né rassegnata. Un anacronismo amorale - se mi permette la battuta - sembra essere il *sentiment* di quel cartello di aziende che, già favorite per decenni da un'assurda secretazione dei contratti di fornitura, fino a tre mesi fa lo erano anche dalla procedura che imponeva di bandire gare per il solo vitto; un appalto che, tuttavia, portava con sé anche la concessione di un servizio. È fuori di dubbio che quantità, qualità e prezzi del cibo nelle carceri sono stati condizionati a danno dei reclusi dall'avidità smodata di questi privilegiati. Ovviamente a monte c'è una debolezza dell'amministrazione penitenziaria, perché secretazione dei contratti, prestazione congiunta di vitto ed extra vitto, aggiudicazione di gare a dispetto di offerte palesemente anomale - ed è accaduto fino a giugno scorso, nonostante le segnalazioni - sono responsabilità del suo Ministero. Voglio credere, però, anche per l'onestà intellettuale che mi è sembrato di cogliere nella sua risposta, che i recenti interventi del Consiglio di Stato e della Corte dei conti - complice anche la raccomandazione al DAP del garante nazionale dei detenuti intervenuta a metà ottobre - abbiamo dato solo la spinta decisiva a una pubblica amministrazione ormai pronta a imboccare la strada giusta e indisponibile a voltarsi indietro. In altre parole, ora si tratta di tenere il punto, Ministro, di non cedere alle pressioni di chi vorrebbe un regime di perenne *prorogatio*, di fare le gare ponte per i contratti annullati e difenderle davanti ai TAR quando, a fronte di certe impugnazioni temerarie, concedono sospensive; di allargare il numero e promuovere la rotazione delle società fornitrici di derrate alimentari e di coinvolgere anche la grande distribuzione. Dal prossimo anno, poi, si tratterà di bandire gare internazionali e vigilare -soprattutto, ma non solo, laddove uno stesso soggetto si aggiudichi vitto e sopravvitto che non siano i 65.000 clienti fissi della filiera a continuare a pagare il prezzo dell'ennesima pena aggiuntiva senza delitto. Trasparenza e rispetto dei diritti di tutti restano la priorità, l'obiettivo a cui tendere tutti insieme.

che ha sostanzialmente l'intendimento di comprendere quello che il Governo intende fare con la magistratura onoraria. È un tema vecchio e nuovo: vecchio, perché fu una delle prime questioni che sottoponemmo alla sua attenzione quando lei divenne Ministro; nuovo, perché nel frattempo sono intervenuti vari fattori, tra cui anche il rischio più che concreto di una procedura di infrazione da parte dell'Europa, stante una sentenza della Corte di giustizia europea che ha puntualizzato alcuni aspetti, a cominciare da quelli del diritto che spetterebbe alla magistratura onoraria in termini di lavoro a termine e, soprattutto, con riferimento a tutta una serie di tutele delle quali oggi è sprovvista.

di condividere lo stato delle attività su questo articolato capitolo della magistratura onoraria. Proprio in questi giorni e in queste settimane sono in corso importanti interlocuzioni tra il Ministero e gli uffici della Commissione europea per risolvere il capitolo più urgente, che è quello delle problematiche relative alle tutele della magistratura onoraria in servizio allo stato attuale.

La Commissione europea ci ha dato degli indicatori ben precisi da seguire e che stiamo effettivamente tenendo presenti nell'elaborazione di una proposta normativa. Per parte nostra, abbiamo un'ipotesi già abbastanza elaborata e stiamo svolgendo i dovuti confronti con tutti i soggetti coinvolti: la Commissione europea, per comprendere se soddisfa le loro richieste, e - parallelamente e necessariamente - il Consiglio superiore della magistratura, per verificare vincoli costituzionali e ordinamentali che condizionano le scelte possibili, le esigenze di funzionalità dei servizi e tutto quello che, in questo momento, ruota intorno al mondo della giustizia. Vorrei sottolineare un punto. Si tratta di un intervento indispensabile per assicurare le tutele dovute ai magistrati onorari in qualità di lavoratori, come richiesto dall'Unione europea. Pertanto, si tratta di un intervento che costa. Penso che l'imminente disegno di legge di bilancio debba tenere conto di ciò e prevedere le risorse necessarie a questo scopo. Realizzare l'esigenza di una disciplina compiuta dello *status* di magistrato onorario in funzione dell'efficienza del sistema giustizia deve necessariamente accompagnarsi allo stanziamento delle risorse

che nelle numerose interlocuzioni intercorse hanno mostrato disponibilità ad accompagnare con gradualità la piena implementazione dell'intervento normativo che stiamo elaborando, il quale è necessario e ormai improcrastinabile. Naturalmente dopo questo intervento sullo stato esistente occorrerà proseguire su tutti gli altri aspetti, sui quali adesso non mi soffermo, pensando al nuovo e a dare attuazione anche alla sentenza della Corte costituzionale

signor Ministro, il Gruppo è sicuramente soddisfatto della risposta che lei ha dato, perché intanto enuclea le tempistiche che supponevamo fossero legate alle problematiche dei costi, oltre naturalmente all'interlocuzione con la Commissione europea. Accogliamo con piacere il fatto che però si parla di legge di bilancio, il che significa tener fede all'ultima proroga che è stata fatta, quella relativa al 31 dicembre, almeno per le situazioni più emergenziali. Abbiamo notato infatti che la questione era stata anche inserita fra i provvedimenti collegati quando è stata fatta la Nota di aggiornamento al DEF. Siamo soddisfatti anche perché ci sembra che sia centrato il punto, cioè l'intervento indispensabile dal punto di vista della qualità del lavoro prestato. Possiamo quindi dire che attendiamo il testo normativo;

Signor Presidente, signor Ministro, premesso che l'articolo 27 della Costituzione dispone che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano tendere quindi alla rieducazione e risocializzazione del condannato, il carcere non è luogo di repressione ma di ordine, sicurezza e trattamento, dove i detenuti sono condotti all'interiorizzazione delle norme, alla responsabilizzazione e al rispetto delle regole, mediante un processo di inclusione fatto di autonomia, socializzazione e integrazione. L'emergenza carceraria legata al sovraffollamento è un problema atavico e consolidato nel tempo, che rischia di compromettere gli ambiziosi obiettivi costituzionali. Innumerevoli fatti di cronaca vedono indistintamente coinvolti detenuti e personale che, a seconda dei casi, risultano presunti autori o vittime di fatti illeciti. Ciò è manifestazione evidente delle inadeguate condizioni di vivibilità per tutti coloro che ruotano attorno alle strutture penitenziarie. mancanza di personale di polizia penitenziaria, di figure trattamentali come gli educatori (vi è una media di circa due per istituto), di dirigenti penitenziari, non solo al Nord ma anche al Sud, tenendo tra l'altro presenti anche i frequenti pensionamenti e l'età avanzata del personale del Sud. Si consideri che risultano essere state riaperte durante il periodo del *lockdown* anche strutture chiuse per inagibilità, esempio una sezione della casa circondariale di Trani, e che risultano essere ancora attivi spacci o bar dove è impiegato personale di polizia penitenziaria, distolto dai suoi precipui

la necessità che gli istituti penitenziari siano dotati di strumenti di controllo automatizzati e che possano essere utilizzati i droni. Molti soggetti che sono privati della libertà presentano patologie psichiatriche e purtroppo bisogna prendere atto che non sempre ci sono delle adeguate articolazioni ASL per la salute mentale.

scorso, e quindi soggetti che transitano *sine titulo* nelle carceri. Per questi motivi, chiedo di sapere dal signor Ministro se sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda intraprendere.

sono numerose, tutte di estrema rilevanza e frutto di problemi irrisolti da molto tempo. Certamente, anche qui, in tre minuti non sarà possibile esporre tutte le attività che, su vari fronti, si stanno approntando per affrontare tutte queste emergenze, tenendo presente sempre quel faro rappresentato dall'articolo 27 della Costituzione. Anzitutto, il problema del sovraffollamento, che lei ha citato, è un problema che persiste nelle nostre carceri. È importante aprire gli occhi su questo fatto. Ho già detto, in più di un'occasione, che è un problema che va affrontato da diverse angolature, ad esempio valorizzando l'esecuzione penale di comunità, con le sanzioni e l'esecuzione della pena diverse dal carcere, l'esecuzione penale esterna, ma naturalmente anche facendosi carico e intervenendo sulle strutture. Ha ragione, senatrice che gli spazi detentivi gravano sulla condizione della detenzione e della vita dei detenuti, ma anche di chi lavora in quelle carceri. È per questo che si sta intervenendo con molte ristrutturazioni, utilizzando tutti i poteri anche acceleratori che sono dati all'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2022 e con i fondi del PNRR, o meglio nell'ambito di quelli complementari: è prevista la costruzione di nuovi padiglioni, di cui mi preme sottolineare che l'intervento riguarda non solo i posti letto disponibili, cioè le camere, ma anche le aree trattamentali. È sempre importante che si portino avanti, soprattutto nei nuovi progetti, degli sviluppi equilibrati. Il personale è in grave carenza e in grave sofferenza. Una delle prime cose che ho fatto, come Ministro, è stato riattivare i concorsi che erano stati congelati durante il periodo della pandemia. Ho chiesto all'amministrazione penitenziaria di pianificare i concorsi con regolarità e con cadenza annuale e, proprio in queste ore, c'è una trattativa del comparto sicurezza per ottenere un ampliamento delle piante organiche. Mi auguro che il Governo e il Parlamento, sempre nella manovra di bilancio, tengano conto di queste drammatiche esigenze. Sulla videosorveglianza fissa, attraverso *bodycam*, videoregistrazione e sistemi antidroni, è da settimane che, soprattutto in seguito a fatti di grave attualità, ho sollecitato l'amministrazione penitenziaria a farsene carico e ci stiamo lavorando. Infine, vorrei fare un accenno al problema della malattia psichiatrica, delle REMS e soprattutto dei detenuti *sine titulo*. Voi sapete che questa è una competenza che è prevalentemente in capo al Ministero della salute, ma non dico questo per esimermi dalle mie responsabilità. Al contrario, abbiamo fatto un tavolo, soprattutto sul finire dell'estate, per cominciare ad affrontare in modo più sistematico questo problema. Le do qualche elemento. Se al 28 ottobre 2020 i detenuti irregolari per malattia psichiatrica erano 98, oggi sono 35. Ancora troppi, ma il lavoro che si sta facendo è molto, con il contributo di tutti, Ministero della salute e Regioni, che in questi mesi sono state sensibilizzate e ci hanno dato la disponibilità di nuove strutture che stiamo attivando. Abbiamo anche l'occhio della Corte costituzionale e stiamo rispondendo, col Ministero della salute, a un'istruttoria richiesta dalla Corte su questo punto. Vi sono problemi di varia natura, anche nel riparto di competenze, perché, ovviamente una chiarezza delle competenze può aiutare una migliore facilitazione nella risoluzione dei problemi.

*(M5S)*. Signor Presidente, oggi la comunità di Portici, Comune della provincia di Napoli, si stringerà nel dolore, nel silenzio e nella preghiera, perché si svolgeranno i funerali di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani di ventisei e ventisette anni uccisi a colpi di pistola tra la notte di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre.

Presidente, in riferimento a questo voglio fare una riflessione. Questa persona deteneva, seppur legalmente, delle armi da fuoco. Faccio mio l'appello di Libera-sezione Campania, in particolare del coordinatore della Provincia di Napoli, il dottor Leandro Limoccia, che faceva delle osservazioni partendo ovviamente da un dato: soprattutto in questa società bisogno di un nuovo umanesimo e quindi di fare in modo che ci siano sempre meno modalità aggressive anche di proporsi al pubblico, alla gente, perché a volte anche le parole pesano. Egli proponeva addirittura di togliere la possibilità di possedere armi da fuoco e quantomeno di agire

perché la persona che ha ucciso questi ragazzi deteneva delle armi e, a suo dire, aveva paura di essere derubata. Questo mostra